lumi, informazioni, approfondimenti, certezze sui dati connessi al concordato fiscale, che ieri è scaduto. Siccome è un punto centrale del confronto che sta partendo sulla manovra e il Governo, in momenti diversi, ha dichiarato che sarebbero entrati 3 miliardi, poi 2, poi temiamo che sia accaduto quello che avevamo paventato. Vorremmo che il ministro Giorgetti rispondesse all'interrogazione della senatrice Tajani. Da quello che leggiamo oggi sui giornali e dalle informazioni che ci arrivano, dovrebbero aver aderito da 150 a 200.000 contribuenti, presidente Malan, su una platea di 4,7 milioni di contribuenti potenziali, di cui 2,7 milioni con pagella fiscale e 2 milioni forfettari. Lo diciamo perché è evidente

un piccolo acconto subito; mentre tutti coloro che sono in difficoltà, coloro che non hanno bisogno di aderire a un condono ovviamente non avranno aderito. Questo ci preoccupa e pertanto la richiesta alla Presidenza è di sollecitare il ministro Giorgetti a rispondere alla senatrice Tajani, che penso possa aiutarci tutti a far luce sulle risorse effettive di questa operazione, che avete definito di *compliance* e che altro non è

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi e colleghe, le Province autonome di Bolzano e di Trento, grazie alla loro autonomia, hanno potuto inaugurare le loro politiche per la montagna più di settant'anni fa con misure contro lo spopolamento a favore dei piccoli Comuni, per il presidio del territorio e per tenere in vita tutta la rete dei masi. Questi temi così importanti sono oggi al centro del provvedimento che stiamo per approvare e rappresentano un contributo significativo per la vita di montagna. Riconosciamo quindi l'impegno e la sensibilità del Governo su questi temi, e in particolare desidero ringraziare il ministro Calderoli e la relatrice Pirovano, che hanno seguito con grande attenzione e con spirito di collaborazione tutto il lavoro parlamentare. La montagna - come il nostro caso dimostra - va affrontata tenendo conto delle sue particolarità, ma anche delle sue continue trasformazioni e delle sue continue sfide. E questo è ancora più vero oggi: innanzitutto vi è la crisi demografica che - come abbiamo visto - ha segnato un nuovo *record* negativo delle nascite; essa avrà le principali ripercussioni proprio sulle aree interne e sui territori di montagna. Già oggi in molti Comuni si fa una gran fatica a tenere in piedi anche i servizi primari. è il cambiamento climatico, che sta trasformando e trasformerà sempre più il modo di abitare la montagna: si avranno più pericoli legati allo scioglimento dei ghiacciai, la perdita di biodiversità, la progressiva erosione dei pascoli.

In questo contesto, una delle più grandi preoccupazioni di chi vive nelle zone di montagna è la crescente presenza dei grandi carnivori, che si inserisce nel complesso panorama delle sfide legate alla gestione degli ecosistemi montani. Domenica scorsa, in un *referendum* consultivo in tredici Comuni della Val di Sole sulla presenza di orsi lupi, il 98,5 per cento dei votanti si è espressa per le politiche più efficaci di contenimento della loro presenza. Questa percentuale dimostra che il tema non è più rinviabile e, pertanto, ringrazio l'Assemblea per aver approvato il nostro emendamento, con cui si compie un primo passo verso il riequilibrio della presenza dei grandi carnivori, in un'ottica di tutela della pubblica incolumità non solo della popolazione ma anche degli animali da allevamento. Per tutte le ragioni espresse e per il fatto che il provvedimento ha il merito di guardare alla montagna come un sistema unitario, che è quello che noi diciamo e chiediamo da sempre, annuncio il voto favorevole dei componenti SVP del Gruppo Per le Autonomie e l'astensione degli altri componenti.

piste della mia terra in Val Senales. Purtroppo la montagna non è solo una bellissima cartolina; va amata e perciò rispettata e temuta, nel suo insieme dell'ecosistema. Solo sulle piste vi sono 30.000 incidenti l'anno, si contano 1.500 ricoveri e 20 decessi, uno ogni 1.700 sinistri; ma nessuno, dico nessuno, si sogna giustamente di chiudere le piste o vietare gli sci. Vorrei che lo stesso atteggiamento, signor Ministro, si avesse nei confronti della fauna selvatica che popola le nostre montagne, e lo dico con cuore e sincerità. Voglio premettere che le mie parole sono figlie di quello sguardo, il mio a 360 gradi per giorni, su un territorio montano tanto vasto, bellissimo e altrettanto complicato, come il mio Trentino-Alto Adige, dove ben il 100 per cento dei Comuni è classificato come montano. Ed è così pure per la Val d'Aosta e per altre Regioni d'Italia, dove le percentuali sono decisamente notevoli. L'Italia L'Italia è costituita in gran parte di aree montuose: parliamo del 49 per cento del territorio nazionale, con oltre 9 milioni di italiani residenti. Per questo mi sono sempre battuta contro lo spopolamento delle zone montane, di cui la mia Provincia, l'Alto Adige-Südtirol, è maestra. E lo è un po' meno paradossalmente invece il Trentino, che è sempre Provincia autonoma, ma dove purtroppo il fenomeno dello spopolamento è invece vigente. È un tema oggi acclarato in tutta Europa e anche per il nostro Paese sta diventando una vera emergenza. Non si tratta più di una fuga, come negli anni Cinquanta e Sessanta. Oggi nei 3.500 Comuni montani

e spesso mancano, nei territori montani, infrastrutture adeguate alle comunicazioni digitali e ancora addirittura telefoniche. Alla fragilità del territorio si aggiungono fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e incendi boschivi. Eppure le nostre montagne sono preziosi custodi di ingenti risorse naturalistico-ambientali, che garantiscono servizi ecosistemici essenziali per l'intero territorio nazionale, a partire dall'acqua e dall'energia elettrica (il 71,7 per cento degli impianti idroelettrici si trova nei Comuni montani). Non si fatica quindi a comprendere il valore, anche in termini economici, delle aree montane, dato che questo territorio non è più il luogo tradizionale del taglio del bosco e non ha soltanto una vocazione agricola, ma aspira ad essere punto di riferimento per l'erogazione dei servizi ecosistemici e per il mondo produttivo, nonostante politiche pubbliche che finora non sono state in grado

e carente rispetto alla rilevanza strategica attribuita anche dalle politiche di sviluppo dell'Unione europea alle aree interne, rurali e montane. Al Sud come al Nord, al Centro e nelle isole aumentano le differenze e le disuguaglianze tra centri urbani e zone montane e gli indicatori demografici ed economici sono concordi nel dire che non c'era altro tempo da perdere per intervenire. E per questo la ringraziamo, signor Ministro. In questi due anni il Governo Meloni ha orgogliosamente raccolto il testimone ormai ingiallito da decenni di generale disinteresse verso la montagna e lo ha fatto impostando un'azione politica seria, mirata e orientata ai bisogni effettivi delle persone che risiedono nelle aree interne e che qui intendono investire. Un provvedimento chiaro,

particolarmente sentito anche nel mio collegio, il Trentino, in condizioni di effettiva parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale. Non a caso all'articolo 3 si parla di strategia nazionale per la montagna italiana. Vogliamo, in altri termini, dare vero valore alla scelta di coloro che intendono restare o tornare a vivere nelle aree interne e dare loro supporto e servizi, garantendo così, al tempo stesso, la lotta al processo di spopolamento con la tutela dell'ecosistema ambientale, perché chi vive e chi fa impresa in tali luoghi possa godere di alcuni importanti vantaggi in grado di riequilibrare le differenze con il resto del Paese. Con questo provvedimento stiamo parlando di misure che possono attrarre maggiori investimenti; di agevolazioni fiscali ed emolumenti speciali che potranno consentire, ad esempio, di dare supporto alla creatività imprenditoriale locale, di attrarre e mantenere operatori nei settori essenziali della scuola e della sanità (più medici e infermieri, così come più maestri nelle nostre vallate). Stiamo parlando di misure che possano creare nuove professioni della montagna, far rivivere borghi incantati, dove la longevità è garantita, e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, la digitalizzazione dei territori e la geolocalizzazione, locale e globale. Stiamo parlando di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e turistico delle nostre zone un obiettivo ambizioso, che però non ci spaventa, abituati come siamo a raccogliere le sfide e ad ascoltare i bisogni che la nostra gente ci affida. Non a caso tutti gli indici di gradimento verso l'azione di questo Governo di centrodestra parlano chiaro, caro collega Boccia, anche attraverso le parole del presidente Mattarella. Questo provvedimento è pensato anche per le giovani generazioni, a cui vogliamo rivolgerci con grande attenzione e cura; le giovani coppie per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa o per i giovani imprenditori. Diverse, infatti, sono le misure agevolative previste e i crediti di imposta perché possano essere incoraggiati a investire, insediarsi e restare in montagna, scongiurando l'abbandono di luoghi e comunità che costituiscono un patrimonio prezioso per il nostro Paese, e magari anche di non abbandonarlo alle mafie. La loro bellezza, il paesaggio, la storia, la cultura e le loro tradizioni linguistiche costituiscono anche geograficamente la spina dorsale della nostra Nazione. Questo testo vuole di certo costituire non il punto di arrivo, ma semmai il punto di partenza per ridare quella doverosa dignità dignità ai territori montani e ristabilire quel minimo comune denominatore con il resto dei territori della nostra penisola. Sarebbe stato bello fosse stato condiviso in queste Aule, perché riteniamo che la strategia nazionale per le aree interne debba essere una strategia comune tra tutti gli attori istituzionali, fondata sulla collaborazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze del sistema Stato e autonomie. Non è più tempo di nascondersi dietro il rimpallo delle competenze: ci sono interi territori che reclamano attenzione, cura e sviluppo. Vogliamo forse aspettare che intere Province dei nostri Appennini restino terra di nessuno? Colleghi, solo chi non vive certe realtà non può comprendere le ripercussioni legate all'abbandono di quelle aree, che sono infatti molteplici, compreso il venir meno della cura del paesaggio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, con le conseguenze alle quali tutti stiamo assistendo, oltre che del tessuto storico-culturale. La risposta allora non può che essere sviluppo, occupazione, attrattività, presenza dell'uomo. Mi riferisco allora in particolare a quelle misure contenute nel disegno di legge rivolte, ad esempio, alle imprese agricole di nuova costituzione, perché possano essere incrementate le attività di promozione e la creazione di relazioni di filiera e di interfiliera nell'ottica di creare dei veri e propri distretti rurali e agroalimentari che possano sviluppare politiche strategiche per la formazione la valorizzazione dei distretti del cibo, rilanciando le produzioni agroalimentari e non. Pensiamo inoltre al turismo rurale che, negli ultimi anni, ha fatto registrare cifre altamente positive. Condividiamo il grande lavoro svolto dal ministro Calderoli, perché dalla residenza dei borghi storici possa anche passare la riscoperta delle produzioni locali. Parchi, beni ambientali, dimore storiche, cammini e ciclovie, che sono patrimonio naturalistico di assoluto spessore, potranno quindi diventare volano di sviluppo per quelle aree interne che fino ad oggi sono state considerate come figlie di un dio minore. Valorizzare le specificità territoriali è un obiettivo non solo possibile, ma anche strategico, che ha nelle diversità territoriali,

per rilanciare l'intero Paese e per questo lo sosteniamo con grandissima convinzione. Benvenuti. Signora Presidente, conservatorismo compassionevole: potremmo rispolverare questo concetto in voga, inventato dai dai repubblicani americani a metà degli anni Settanta e diventato il pilastro ideologico, concettuale e culturale su cui Bush padre e, in particolare, Bush figlio costruirono le loro politiche negli Stati Uniti d'America. È l'idea, cioè, che nei confronti dei territori, delle realtà più disagiate e, più in generale, sulle esigenze degli interventi nel campo del *welfare*, lo Stato non dovesse dare delle risposte di natura organica per andare a rimuovere le cause e le condizioni del disagio e della diseguaglianza, ma dovesse tutt'al più donare qualche mancetta, qualche previdenza, qualche beneficenza, atta perlopiù ad evitare che chi è in condizioni di difficoltà disturbi il manovratore. Ecco, se vogliamo avere una rappresentazione plastica di questa concezione, di questa idea, di questa politica, possiamo tranquillamente prendere prendere in mano questa legge: è conservatorismo compassionevole, che unisce un'impostazione di impronta sostanzialmente individualista, demolendo intimamente un'idea profondamente identitaria nei territori montani, che è l'idea comunitaria, è l'idea autonomistica, trasferendo su questo impianto sostanzialmente individualista (ciascuno basti e pensi a sé) una impostazione di natura statalista, che però frana inevitabilmente nel momento in cui si presume di passare all'incasso. Poco fa, in quest'Aula, ho sentito una descrizione irenica. irenica. Ma mi spiegate come sia realmente possibile realizzare quel Paese dei campanelli - qualcuno qui lo ha definito con la stratosferica, fantasmagorica, incredibile cifra di 100 milioni di euro all'anno, che dovrebbero coprire tutte le misure - in una dimensione nella quale quale voi avete fissato strettamente i binari della finanza pubblica e mantenendo questo impianto dentro una dimensione di trasferimenti statali, cioè di finanza derivata?

perché aveva mantenuto un impianto di finanza derivata come lo mantiene oggi. E, quando in quel momento arrivò una congiuntura economica negativa, con i tagli lineari si andò a pescare laddove si doveva e poteva andare a pescare. E lo si fece addirittura, allora, mettendo in piedi una demagogica campagna nei confronti degli enti che governano questi territori che portò alla demolizione, alla distruzione, al depauperamento del tessuto istituzionale montano nel nostro Paese. Lo avete fatto voi e adesso venite qui a farci la morale, a risciacquarci la coscienza dicendo che state salvando questi territori? Un minimo di pudore servirebbe, se non necessariamente e propriamente un minimo di memoria. Ma veniamo alla questione di fondo. Colleghi, la montagna italiana oggi è il grande malato di questo Paese, perché anticipa dinamiche che colpiranno l'intero Paese se non ci saranno delle politiche adeguate di risposta. Oggi in quei territori due persone escono dal mercato del lavoro e, quando va bene, una ne entra. Quindi, si pone un problema drammatico di sostenibilità del *welfare* e dello Stato assistenziale, perché in quei territori l'inverno demografico è molto più accentuato che nel resto del Paese, perché la fuga dei giovani è più accelerata rispetto al resto del Paese. Cari colleghi, se in dieci anni 550.000 giovani se ne sono andati da questo Paese, forse dovremmo interrogarci tutti. Mentre noi facciamo polemiche sulle questioni futili, stiamo perdendo l'impianto del futuro su cui dovremmo costruire il nostro avvenire. *(Applausi)*. In quei territori è in atto una dinamica che pare inarrestabile, che va sotto la voce di spopolamento.

e quel tema non è che non ci riguardi, purtroppo - l'abbandono dei terreni, lo sfruttamento di risorse naturali ai fini produttivi - penso al tema dell'energia verde - che utilizzano acqua, suolo, foreste, vento, in una dinamica in cui i territori vengono espropriati della capacità di intervenire. Quei territori hanno un tessuto amministrativo in crisi,

di fondo sui livelli istituzionali. In sostanza, tale quadro avrebbe richiesto una proposta organica, che invece non c'è. Come ho detto, siamo in presenza di una norma manifesto, buona per i *like* sui *social* che può essere utilizzata nei comizi a facile presa, ma che sarà - è facile essere profeti in questo senso - totalmente inefficace per fornire le risposte in grado di invertire la dinamica. Con

che si presenta nelle Aule parlamentari per sostenere le ragioni del Mezzogiorno. Faccio presente che con l'articolo 2 il Mezzogiorno sarà particolarmente colpito, perché si interverrà sulla classificazione dei Comuni montani escludendo pezzi significativi e interi dell'Appennino e delle isole. Capisco che adesso bisogna seguire la nuova linea del compagno Travaglio, che dice che siete pronti a entrare nella nuova maggioranza di Governo con la destra. Tuttavia, venire qui a fare la morale sulle politiche del Mezzogiorno e poi non votare contro questa misura - è contro contro il Sud e le aree disagiate interne del Mezzogiorno e aumenterà ed enfatizzerà le diseguaglianze - significa essere sostanzialmente dei sepolcri imbiancati.

statalista, con lo Stato che interviene su elementi che hanno bisogno di una loro capillarità profonda. E invece non l'avete fatta, perché siete divisi. Siete divisi fra di voi: tra chi vuole reintrodurre le Province a elezione diretta, chi vuole fondere i piccoli Comuni e chi vuole l'autonomia differenziata. Dentro questo *bailamme* non fate nulla perché i soldi non ci sono e, quindi, rinviate. Le riforme si faranno sempre domani e così i territori arrancheranno. Il secondo perno della questione per lo sviluppo di questi territori, che noi abbiamo cercato di portare all'interno delle proposte emendative, ma voi avete chiuso, è il tema di come si garantiscono salute, trasporti, scuola e assistenza, che sono elementi fondamentali. La terza e ultima questione è il tema di come si fa sviluppo locale, di come le comunità locali vengono messe nelle condizioni di poter utilizzare le risorse di quei territori per generare reddito, occupazione, sviluppo e ricchezza. ricchezza. Signora Presidente, questa è una legge da Statuto Albertino che, a metà fra grida manzoniane e soluzioni velleitarie, ci riporta indietro. Si pensi, ad esempio, alla questione relativa all'articolo 24. La *premier* Meloni ci ha detto basta *bonus*. Qui pensate di dare una mancetta di 50 euro - ripeto, 50 euro - a chi avrà un bambino in quei territori. la cifra molto chiara della rappresentazione del fallimento di questo tipo di impostazione. Per tutto quanto esposto, non siamo favorevoli e non comprendiamo il motivo per il quale altri, invece, avalleranno un'impostazione di tale natura.

la deludente proposta che va in questa direzione. Intanto vorrei sottolineare, ad esempio, che in 5a Commissione

Il Ministro lo sa. Voglio ragionare su questi temi: in quel Comune una coppia giovane di fatto non può andare

problema dei trasporti. Quanto costa, ad esempio, la questione del trasporto? Ecco, una volta tanto proviamo a discutere concretamente della vita che vivono le persone, altrimenti

Non potete venderlo come un'inversione di tendenza, nel senso che non dà risposte in questa direzione, perché - lo ripeto - le risorse sono insufficienti e, allo stesso tempo, non si aggrediscono alcune caratteristiche.

Signor Presidente, gentile Ministro, innanzitutto ci tengo a ringraziare il Ministro, la relatrice Pirovano e il presidente Balboni, anche se non è in Aula,

un testo non solo adottato in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, che prevede la valorizzazione delle zone montane, ma che intende anche migliorare l'amministrazione e l'attrattività di quei territori. Parliamo di 3.524 Comuni montani, cui si aggiungono altri 652 parzialmente montani. In termini di estensione, questi rappresentano quasi la metà di tutto il territorio nazionale. ho detto e come hanno ricordato in tanti, la legge vigente che riguarda la montagna ha ormai trent'anni. Con questo nuovo testo si intende definire in modo organico le politiche destinate ai territori montani, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. All'interno del quadro delle competenze, oltre allo Stato, ogni ente del territorio adotta gli interventi necessari per lo sviluppo socioeconomico, la tutela e la valorizzazione della specificità delle zone montane. Nell'ambito dell'esame in Commissione sono state approvate diverse proposte di Forza Italia. specifica che gli interventi da parte dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome debbano essere adottati mirando a una risposta perequativa, finalizzata alla rimozione delle diseguaglianze derivanti dallo svantaggio economico e sociale delle zone montane. È previsto che siano stabiliti i criteri per una puntuale classificazione dei Comuni che costituiscono le zone montane, quindi viene definita la strategia nazionale per la montagna italiana, disponendo, in merito alle modalità di finanziamento, degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Ci si pone quindi il tema di valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture che sono nei Comuni montani. A loro sono destinate misure di sostegno, come un credito di imposta per la locazione a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie di montagna o vi effettuano il servizio medico, cioè per tutti quei medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale. Un analogo sostegno è destinato anche al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo. Un altro emendamento accolto, sempre di Forza Italia, prevede l'estensione, a tutti i Comuni montani nei contesti di disagio giovanile o caratterizzati dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, della deroga al numero minimo di alunni per classe con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e percorsi sperimentali nella scuola secondaria di secondo grado. Questa misura si aggiunge alle disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane, prevedendo la possibilità, per le università e le istituzioni di aventi ovviamente sede nei territori dei Comuni montani, di stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane. Al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali in quelle aree, vengono previsti i contratti di programma per le concessioni della rete stradale e ferroviaria, con specifici interventi sulle infrastrutture, ovviamente, di rispettiva competenza. Abbiamo anche proposto che, tra le priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, vi sia la rimozione delle barriere che limitano la copertura dell'accesso alla rete in banda ultra larga e l'eliminazione del divario digitale. Un ulteriore emendamento di Forza Italia immagina che la strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani preveda il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle diverse amministrazioni, anche dagli enti locali. Tra i servizi da rendere, ovviamente ce n'è un altro importantissimo, che è quello della telemedicina, ma si punta anche all'attivazione ed all'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati, nei quali erogare ovviamente servizi in presenza, con particolare riferimento ai Comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento. Vi è inoltre il tema dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione e della certificazione delle foreste e della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati. Una modifica inserita nel testo su nostra proposta introduce il concetto di agricoltura di montagna per la sua valenza multifunzionale di presidio antropico, ambientale ed economico. In questo modo, si riconoscono quelle montane come zone florofaunistiche a sé, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali. Inoltre, nel testo c'è la previsione di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane, attraverso attività di monitoraggio dei ghiacciai, nonché attraverso la realizzazione di casse di espansione, vasche di laminazione e bacini idrici. Con una nostra proposta, ora nel testo, sarà possibile l'utilizzo idroelettrico nel novero delle azioni attuabili per prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica. Ciò crea il presupposto per un eventuale futuro accesso al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, che sostiene interventi a carattere straordinario. Sono inoltre previsti incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori di montagna. Viene introdotta una definizione di rifugi di montagna, lasciando alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di stabilirne le caratteristiche funzionali. A riconoscimento delle professioni della montagna, viene data loro importanza quali fondamentali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, mentre per le imprese esercitate da giovani sono previste apposite misure di agevolazione fiscale. Inoltre, viene individuato uno sgravio contributivo per agevolare il lavoro agile nei Comuni montani con meno di 5.000 abitanti: è una misura per i lavoratori giovani che trasferiscono in uno di questi Comuni l'abitazione principale e il domicilio stabile. A tal fine è previsto pure un credito d'imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale. Insomma, andiamo verso una nuova legge per la montagna che, oltre a riconoscere il valore delle zone montane, mette in campo disposizioni pratiche e di agevolazione fiscale per ridurre la distanza tra la montagna e la città. Per queste ragioni, annuncio il voto convintamente favorevole dei senatori di Forza Italia. Presidente, siamo tutti d'accordo sul fatto che si debba lavorare per la promozione delle zone montane e questo provvedimento, almeno dal titolo, sembra andare in questa direzione. in esame è pieno di buone intenzioni e di buoni propositi; peccato però che a remare contro sia proprio il Governo, quando si tratta di definire le risorse economiche da mettere in campo. Colleghi, non so se ve ne rendete conto, ma con 200 milioni di euro pensate di sistemare i problemi relativi alla sanità, all'istruzione, alle infrastrutture tecnologiche e ai sistemi di trasporto e di creare opportunità di lavoro su una platea di 4.000 Comuni, che sono più o meno mezza Italia, come ci diceva prima la collega Ternullo. Ternullo. Colleghi, gli obiettivi sono ambiziosi e noi li condividiamo, ma il Governo sta limitando fortemente le risorse da destinare a questo provvedimento e, allo stesso tempo, non si fa scrupoli a spendere 680 milioni di euro per un terreno in Albania, facendo finta di aver risolto il problema dell'immigrazione. Colleghi, voi state spendendo i soldi degli italiani per fare propaganda elettorale e poi ci venite a dire che non avete i soldi. La cosa più grave è che voi adesso state continuando a dire che la colpa è dei Governi che vi hanno preceduto. Non rendetevi ridicoli: siete già arrivati alla terza legge di bilancio e ancora è colpa dei Governi che vi hanno preceduto?

State dimostrando di non capire neppure la differenza che c'è tra gli sprechi che fate voi e le misure di rilancio dell'economia che abbiamo fatto noi, quando eravamo al Governo. Ci fate capire che non vi interessa nulla dello spreco di denaro pubblico, perché non volete neppure combattere con quell'enorme spreco di denaro pubblico che si chiama corruzione, che costa 237 miliardi l'anno all'Italia. Non lo fate perché, anziché combattere la corruzione, state combattendo contro le procure e contro la magistratura. Il problema non è soltanto il fatto che non mettete risorse economiche. Quello che manca in questo provvedimento è la visione sul futuro economico da dare alle aree montane. Qual è il vostro progetto per il futuro di queste aree? Al di là delle parole che state inserendo in questo provvedimento, cos'è cos'è che manca? La grande assente in questo provvedimento è una strategia credibile per il futuro di queste aree. Volete valorizzare ad esempio la vocazione turistica? Allora pensate di fare dei comprensori, magari di sport di montagna, ma servono investimenti massicci. Come pensate, con questa elemosina, di rilanciare l'economia delle zone montane? E perché dovremmo fidarci di questo Governo, quando già state dimostrando, nella ricostruzione del Centro Italia, di non essere in grado di capire che non basta ricostruire le case, se non si investe nel futuro economico e nello sviluppo economico di questi paesi? C'è però un'altra preoccupazione che non posso tacere. Questo Governo adesso si riserverà di definire i criteri per stabilire non tanto quelli che saranno "Comuni montani", ma quelli che non lo saranno più.

se questo provvedimento, una volta che avrete definito il suddetto criterio, si chiamerà ancora "zone montane" oppure si chiamerà "zone alpine". Questo ancora non ci è chiaro, perché, a quanto pare, saranno penalizzate proprio le Regioni del Centro-Sud.

quando si parla alle nuove generazioni, dobbiamo prestare molta attenzione a non vendere illusioni. Io mi preoccupo, perché questo Governo purtroppo è abituato a vendere illusioni. Avete venduto illusioni ai vostri elettori quando avete parlato di *flat tax*, quando avete parlato di pensioni minime, quando avete parlato delle accise sulla benzina in campagna elettorale. parlato delle accise sulla benzina in campagna elettorale. Avete fatto una campagna elettorale e governate grazie a una strategia di manipolazione che presto gli italiani scopriranno. Presidente, i giovani hanno bisogno di certezze, perché credo che una delle più grandi frustrazioni delle nuove generazioni sia proprio vivere in questo senso di precarietà. E allora non creiamo aspettative che poi saranno disattese. I giovani hanno bisogno di avere la possibilità di costruire un futuro di vita; se non pensate di fare investimenti significativi per la montagna, non create ulteriori illusioni.

che vivono nei territori montani (stiamo parlando di più della metà del territorio italiano). Il nostro sarà un voto di astensione, con l'augurio però che questo Governo abbia almeno un ravvedimento operoso.

nel 1947 il senatore friulano Gortani diceva la politica si ricorda della gente di montagna solo per imporre tributi, redigere norme assurde e prelevare soldati. Membro dell'Assemblea costituente, fu ispiratore dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione ebbe la lungimiranza di considerare le montagne come una realtà da tutelare e difendere; purtroppo però da allora, fatto salvo il prelievo dei soldati, le sue parole risuonano ancora troppo attuali. Era dunque necessario ridare dignità e centralità alle popolazioni delle terre alte, riconoscendo le loro peculiarità e le loro differenze, uscendo dalla logica del mero assistenzialismo. Vivere in montagna è una scelta, un onore e a volte un sacrificio. Nessuno vuole abbandonare la montagna per scelta, ma troppo spesso le persone sono costrette a farlo per necessità ed è qui che dobbiamo intervenire. un provvedimento che non vuole regalare niente a nessuno, ma solo riconoscere le differenze tra aree urbane e montane, sottolineando il valore del lavoro che svolgono i montanari ai fini della tutela e della salvaguardia del territorio, lavoro di cui tutti poi possono beneficiare. Le montagne hanno nel nostro Paese un valore simbolico importante. Vi si radicò la Resistenza durante la Seconda guerra mondiale e da lì nacquero i primi movimenti autonomisti, che già allora videro la prevaricazione della città sulla montagna. Noi vogliamo andare oltre la contrapposizione, ma anche riconoscere a ciascuno il proprio valore. Per la prima volta, il riconoscimento, la promozione, la crescita economica e sociale e il ripopolamento delle zone montane diventano obiettivi di interesse nazionale e lo diventano con una strategia concreta e di amplissima portata, con misure che toccano gli ambiti più disparati. Cito a titolo esemplificativo: misure in materia di sanità, con attribuzione ai fini della valutazione dei titoli in carriera per i concorsi di un punteggio doppio per ogni anno di attività nei Comuni montani; con titoli preferenziali per gli incarichi di direttore sanitario; con contributi sotto forma di credito d'imposta per le locazioni e per l'acquisto di immobili ad uso abitativo, per contenere l'impegno finanziario dovuto al trasferimento; emolumenti di natura accessoria per chi lavora in montagna; misure in materia di scuola, con punteggi aggiuntivi ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza per i docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna; caso, contributi sotto forma di credito d'imposta per le locazioni e l'acquisto di immobili ad uso abitativo; e poi misure per favorire la cultura, la connessione digitale e la mobilità; e ancora, misure per la tutela del territorio attraverso la valorizzazione dei pascoli e dei boschi, dei ghiacciai, dei bacini idrici, dell'agricoltura, della gestione forestale e dei rifugi; misure per l'industria, il commercio, l'artigianato, il turismo e la tutela del patrimonio culturale e montano; per le professioni di montagna, misure fiscali per le imprese esercitate dai giovani, agevolazioni per il lavoro agile, incentivi per l'acquisto e la ristrutturazione delle abitazioni principali in montagna; incentivi per la natalità; registro dei terreni silenti e tanto altro ancora. due parole in più all'articolo 18, frutto di un emendamento da me presentato e del lavoro enorme svolto tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie e quello della giustizia. Il principio introdotto è rivoluzionario, perché modifica le norme in materia di responsabilità; passa infatti il principio che chi va in montagna deve essere consapevole dei rischi che incontra e non si trova in un parco giochi e, nel momento in cui si decide di affrontare la montagna, lo si deve fare a proprio rischio e pericolo. La natura è potente e stupenda, ma per questo anche imprevedibile e pericolosa, e va affrontata con il dovuto rispetto. È assolutamente impossibile mettere in sicurezza un territorio verticale. abbiamo un patrimonio immenso di sentieri e strade poderali da percorrere non solo a piedi, ma anche in bici, soprattutto oggi, con l'esplosione dell'utilizzo delle bici elettriche, che permettono di andare in salita a chiunque. patrimonio viene messo a disposizione dei turisti, che saranno informati dei rischi che affrontano. Come contropartita, con questo articolo oggi si mette un freno alle richieste di risarcimento danni a seguito di sinistri, domande che troppo spesso vengono attivate come se ci si trovasse su una strada di città o su una ciclabile, con enormi ripercussioni sui soggetti che prestano un servizio alla collettività e alla tutela del territorio, mantenendo agibili sentieri e strade poderali. Tutte queste misure sono volte a promuovere la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, rendendoli attrattivi per tornare a viverci e consentendo un effettivo accesso anche a tutti i servizi essenziali. Risorse importantissime verranno finalmente destinate ai Comuni effettivamente montani *(Applausi)*, con criteri che andranno a definire che cosa è montagna davvero e che cosa non lo è. con alcune considerazioni personali. In un mondo che dal mio punto di vista sta diventando sempre più disumano, in cui la vita è diventata sempre più superficiale veloce e in cui i rapporti umani sono sempre più legati al puro apparire, solo la natura ci può salvare. Vivere in montagna, a contatto con la pura bellezza della natura, apre mente e cuore e riporta l'uomo alla sua vera essenza. Questo disegno di legge costituisce uno strumento importante per dare non solo a coloro che hanno avuto l'immenso privilegio di nascere in territori montani di continuare a viverci senza doversene andare, ma soprattutto per dare a tante persone la possibilità di pensare a un cambio radicale di vita trasferendosi in montagna. Le città diventano luoghi sempre più alienanti e sempre più persone in futuro vorranno poter lavorare da una casa a contatto con i boschi, con i figli che possono giocare con altri bambini senza i pericoli del mondo odierno, che costringe tutti a vivere in gabbia. Svegliarsi la mattina riempiendosi gli occhi del colore degli alberi e del cielo, lasciarsi accarezzare la pelle dall'aria pulita e dai profumi intensi ed essere coccolati dal canto degli uccelli non ha prezzo: tocca le corde dell'anima in profondità e sempre più persone in futuro vorranno poter vivere questo. Per tutto questo, porgo un ringraziamento immenso a Roberto Calderoli e alla Lega, perché nell'enorme quantità di provvedimenti di questa legislatura, il disegno di legge autonomia e il disegno di legge montagna, entrambi frutto del lavoro, della determinazione e della capacità del Ministro, sono i due che più mi aprono il cuore. Da fiera valdostana, da fiera autonomista e da fiera montanara, mi inchino e dico grazie, soprattutto perché ho avuto il grande onore di lavorare su entrambi i testi per tanti mesi in 1a Commissione. Ringrazio poi tutta la maggioranza e in particolare i relatori, il presidente Balboni, ma soprattutto un ringraziamento speciale lo porgo alla senatrice Pirovano per l'enorme lavoro svolto. Con orgoglio, quindi, annuncio che il Gruppo Lega voterà a favore del provvedimento. del Governo, ben consapevoli della grande fragilità che caratterizza le aree montane nel nostro Paese, da molto tempo riteniamo necessario un intervento organico e compiuto che se ne faccia carico e senz'altro abbiamo salutato come positivo il fatto che il Governo abbia deciso di occuparsene, presentando

Siamo però chiamati oggi a giudicare il risultato di queste buone intenzioni che il Governo ha proclamato e anche come il Governo, rispetto alle finalità enunciate, che sono condivisibili, ha poi agito sul piano dei mezzi, perché la politica non può mai essere enunciazione di fini senza predisposizione di mezzi adeguati per raggiungerli, altrimenti non è un'attività onesta intellettualmente, ma una presa in giro dei cittadini. Da questo punto di vista, il giudizio che diamo è estremamente critico. Come è stato detto anche da altri colleghi e da tutti i senatori del Gruppo Partito Democratico che sono intervenuti, quella in esame - lo dico senza voler fare polemiche di basso livello è stata presentata come una legge quadro, ma a noi sembra più che altro una legge manifesto, una legge bandiera: non ha le caratteristiche e gli attributi che una seria legge quadro deve avere. In primo luogo, non ha quello che giustifica l'adozione di una legge quadro, e cioè la predisposizione di stanziamenti adeguati che rendano credibili gli impegni che si prendono nei confronti di determinate popolazioni, quelle delle aree montane del nostro Paese, che appunto vivono in condizioni di grande fragilità fragilità e di grande difficoltà, che scontano un accesso ai servizi fondamentali più difficile di quello che c'è in altre parti del Paese e che avrebbero bisogno di scelte più serie, più concrete e meno

la saggezza popolare, un sacco vuoto difficilmente sta in piedi: questa mi pare una buona descrizione del disegno di legge al nostro esame. Dobbiamo

io sono un uomo pratico e devo dire che è meglio qualcosina che niente. Noi non possiamo non essere d'accordo con questo. Il dibattito non può essere sul fatto se qualcosina sia meglio

pronti a convenire. Diciamo però la verità e non inganniamo i cittadini. L'altra incoerenza da sottolineare riguarda il quadro complessivo in cui il provvedimento si colloca. Si mettono 100 milioni in più

alla decisione di tagliare 8.000 posti nella scuola (6.000 per personale docente e 2.000 per il personale ATA)? Cosa sono di fronte alla scelta molto grave di far arrivare il rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL al 6,05 per cento, cioè al livello più basso degli ultimi quindici anni in Italia? Non si può tagliare la sanità a livello nazionale e poi presentare come la madre di tutte le svolte il sostegno ai medici di base nelle aree montane. Questa è un'operazione di contraffazione della realtà che mi pare davvero poco trasparente e intellettualmente credo che si debba mettere l'accento su alcuni forti limiti del provvedimento. Il primo riguarda i criteri per la definizione di Comune montano, che sono troppo restrittivi, oppure errati e lasceranno fuori centinaia di Comuni che invece sarebbero meritevoli di tutela. l'assenza di fondi adeguati, che abbiamo più volte richiamato; la mancata disciplina dei servizi ecosistemici, che è anch'esso un problema di non poco conto; l'assenza di l'assenza di una fiscalità di vantaggio per i Comuni montani, con un rimando alla delega fiscale che è un altro trucco, perché sappiamo tutti che è un fantasma: si mette quindi in campo un fantasma che, per diventare concreto, aspetta che un altro fantasma diventi concreto. Di solito però in questi casi resta solo il fumo e non si vede l'arrosto. Io penso che finirà così anche per la fiscalità di vantaggio per i Comuni. Infine, c'è l'assenza di qualsiasi scelta di riordino degli enti locali. Sul TUEL non abbiamo notizie certe. Lo scenario che abbiamo di fronte è arlecchino e manca un'idea di riordino complessivo del sistema di governo degli enti locali e delle aree montane in particolare. Tutti i nostri emendamenti sono stati bocciati,

estremamente condizionato perché se, come anche hanno chiesto le associazioni dei Comuni montani in queste ore, alla Camera non dovessero essere apportati al provvedimento tutti i correttivi che lo porterebbero al di sopra della soglia di decenza, è chiaro che l'atteggiamento del Partito Democratico, che ora è di dubbiosa, ma responsabile apertura, diventerebbe nell'altra Camera di fortissima contrarietà. Nel dire questo, ci auguriamo quindi che ci possa essere anche una terza lettura al Senato, perché alla Camera ci saranno state modifiche, nella quale saremo in grado di dire al ministro Calderoli, al Governo e alla maggioranza che siamo lieti che le nostre proposte siano state almeno in parte accolte. Il nostro sarà quindi un voto di astensione. Ora però, se la Presidente mi concede altri due minuti, non due parole, anche in sede di dichiarazione di voto, su quello che è avvenuto ieri in Senato e che, secondo me, non è stato messo abbastanza sotto la lente di ingrandimento. Non possiamo abituarci a uno spettacolo come quello che ieri è andato è andato in scena, che, diversamente da quanto è stato detto da alcuni colleghi della maggioranza, non ha precedenti, perché non c'è nessun precedente di un decreto-legge che riguarda un provvedimento pericoloso e controverso, discusso a livello nazionale ed europeo, che è finito sotto la lente di ingrandimento della Corte di giustizia europea, che con uno stratagemma viene sottratto all'esame del Senato, trasformato in un emendamento e portato nell'altra Camera.

il fatto che non era mai successo che si votasse per negare delle audizioni. Si è detto che non si possono fare audizioni su un provvedimento che cambierà:

confronti di queste prepotenze del Governo, che non danneggiano la minoranza parlamentare, ma tutto il Parlamento e non andrebbero lasciate passare.

non solo per come ha gestito, assieme ai due relatori - il senatore Balboni e la senatrice Pirovano - l'*iter* in Commissione, ma anche per aver voluto portare all'attenzione di questo consesso e del ramo più alto del Parlamento una legge sulla montagna all'inizio della legislatura. I toni trionfalistici, quelli sì, che ho visto

gli addetti ai lavori sanno che una legge all'inizio della legislatura ha molte più possibilità di vedere la luce rispetto a una presentata a fine legislatura, ma anche tanti nostri cittadini ormai sono convinti che il pleonastico esercizio delle *boutade* relative alla

concretezza, che è tipica dell'essere montanari. Guardate, io uso questo termine a beneficio di tutti coloro che credono che vi sia un'accezione negativa;

che per scelta del mio partito oggi ha un rappresentante. *(Applausi)*. Infatti, coloro i quali oggi danno lezioni a Fratelli d'Italia e a questo Governo, non hanno espresso o non hanno voluto inserire in posizione eleggibile un rappresentante bellunese e questo già basterebbe per significare l'importanza che ciascuno di noi dà rispetto a taluni temi. In questi taluni temi. In questi due giorni in Assemblea abbiamo sentito, da una parte, l'opposizione parlare di spopolamento. Io ho apprezzato il mio amico e collega Martella quando ha parlato dello spopolamento del mio paese e dei paesi limitrofi. Mi corre l'obbligo di ricordargli, però, che non è un processo che ha visto il suo inizio e la sua maggiore manifestazione durante il Governo Meloni, anzi: è un processo che, anche grazie alle politiche del centrosinistra, si trascina da qualche anno. *(Applausi)*. Ma io non voglio entrare nella polemica tra che lo spopolamento si combatta con le politiche del centrosinistra e chi con quelle del centrodestra, voglio uscire da questo schema; intendo invece cercare di capire se

- a volte eccessiva filosofia, trasformata quasi in lezioncina - di chi cita il Marchese del Grillo, arroventandosi su qualche cavillo della legge, per non dire che quando amministrava nulla ha fatto per la montagna, nonostante ricoprisse ruoli anche straordinariamente importanti. *(Applausi)*. Ma non voglio entrare

che nel giro di vent'anni il 70 per cento della popolazione vivrà in aree urbane e solo il 30 per cento nelle aree rurali. Approfitto per chiedere e cercare di capire se, a dieci anni di distanza dalla legge e dai provvedimenti sulle aree interne, oggi possiamo sentirci soddisfatti di quei provvedimenti. Credo che potrebbe essere oggetto di un'indagine conoscitiva, per capire gli effetti reali di ciò di cui sto parlando, e ritengo che il Parlamento possa e debba interrogarsi su questo. Torno sullo spopolamento per dire che dobbiamo ragionare assieme. Lo dico da ex sindaco, da persona che, in qualche maniera, ragionevolmente, di questi temi si è occupata.

il termine sindrome di Heidi, cioè quel luogo dove «ti sorridono i monti», banalizzando la questione della montagna, facendo credere a milioni di turisti che la montagna sia facilmente accessibile, con i costi che poi gravano, poi gravano, per il recupero in montagna, sia sulle fatiche dei soccorritori del soccorso alpino - a cui credo oggi si debba tributare un grandissimo applauso in quest'Aula sia nei confronti delle risorse che ciascuno di noi mette nella fiscalità, pensando che il mare sia una cosa di cui comunque avere timore, quindi meglio rimanere sulle spiagge, mentre la montagna sia accessibile a tutti, anche con gli infradito. Non è così, è qualcosa di diverso.

per sostenere gli agricoltori e definirli, come il mio amico Bergesio giustamente propone, custodi della montagna. *(Applausi)*. È vero, infatti, che non possiamo pensare che la montagna sia il luna park della pianura, posto che io, se la gente viene in montagna a fare turismo e paga, sono il primo ad essere felice e voglio far crescere la cultura dell'accoglienza nei territori montani. Voglio, però, che sia chiaro che il ruolo del montanaro è anche quello di difesa idrogeologica di questo territorio: non esistono pianure sicure se non esiste montagna sicura; se non esiste la gente che ci vive; se non esistono le risorse destinate a questo bene. Bene ieri ha fatto qualcuno, quando ho citato una percentuale di risorse che dovrebbero essere destinate al dissesto idrogeologico, a ricordare che ci sono, nei canoni idrici, che però qualche Regione ha deciso di destinare anche al funzionamento dell'ente Provincia, dopo che qualcuno quelle province le aveva massacrate e chiuse. Altrimenti dimentichiamo di ricordare che gli assetti del territorio, senatore Parrini, è meglio che non li facciate, perché, quando li avete fatti, avete fatto fare passi indietro a questa Nazione, non passi in avanti. Oggi lo stesso nelle aree locali, anche per bocca dei propri segretari provinciali, si scaglia contro la riforma Delrio: non sono solo voci a favore. Si dimostra così il vostro fallimento, non quello di un Governo che cerca di aggiungere risorse a strategie. Vi dà fastidio. Lo posso capire, Lo posso capire, perché la filosofia della *boutade*, della montagna vista dalla pianura, seduti su un divano, oggi contrasta molto, invece, con una legge che, puntualmente, su sanità, scuole, giovani, *smart working*, agricoltura, pascoli, alberi monumentali, tribunali,

chi c'era prima o chi non c'era prima. *(Applausi).* Il senso di responsabilità con cui amministriamo questa Nazione, infatti, deriva dal fatto che la destra amministra così, anche tanto dal fatto che noi dobbiamo rimediare ai 150 miliardi di debiti che avete fatto su questa Nazione. *(Applausi. Commenti).* Guardate, visto che avete amore nel citare sempre gli enti locali, chiunque abbia amministrato anche solo la cuccia del cane, anche solo la cuccia del cane, sa che nessun Comune avrebbe mai potuto contrarre un debito senza la copertura finanziaria: cosa che voi avete fatto con il superbonus. Vergogna!

il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di cinque articoli. L'articolo 1 prevede che il giorno 24 di ciascun anno sia riconosciuto quale Giornata nazionale delle periferie urbane, al fine di conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di inclusività, sostenibilità e sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale, culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie. Si specifica che tale Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. L'articolo 2 disciplina le L'articolo 2 disciplina le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale, prevedendo in particolare che in tale occasione lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni possano promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti del terzo settore e con

e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini sulle specificità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo. nazionale)* 1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

la prego di attendere un attimo. Chiedo a chi intende lasciare l'Emiciclo di farlo cercando di ridurre il brusìo, in modo che la senatrice Musolino possa intervenire in dichiarazione di voto.

Presidente, ma ti fai rispettare o no? Senatore Scalfarotto, ho già richiamato io. assistiamo spesso a queste situazioni, in cui, durante gli interventi e maggiormente durante le dichiarazioni di voto, il Governo è impegnato in conversazioni con componenti della maggioranza. Ma questo non è rispettoso nei confronti dei parlamentari e dei senatori. E talvolta non è neanche del tutto responsabilità del Governo, perché molto spesso il rappresentante del Governo si trova ad essere assalito dal collega della maggioranza e quindi deve dargli ascolto. Però non è edificante né per chi rappresenta il Governo, né per il parlamentare che deve parlare e deve fare il suo intervento, né per lo spettacolo che viene offerto, sinceramente. A maggior ragione, non è edificante per il senso e il ruolo delle istituzioni che si celebrano in quest'Aula. Quindi mi auguro che vogliamo porre fine a questa pratica. *(Commenti)*. Se poi il mio collega, che in questo momento mi sta riprendendo verbalmente a voce alta, pensa di far cessare il mio intervento

riuscire a terminarli, dobbiamo lasciare il tempo e il modo di intervenire a tutti. MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Grazie, Presidente. Venendo al merito della questione, la Giornata nazionale delle periferie, stavo annunciando il voto di astensione

ma poi ognuno per sé, Dio per tutti e i soldi chissà dove li prendiamo; non è questo il modo per trattare il tema delle periferie. La giornata del 24 giugno viene scelta, evidentemente, per un senso preciso di riferimento a fatti di cronaca terribili e brutali e quindi ci deve richiamare a un rispetto e a un impegno specifico nei confronti delle periferie. I contesti periurbani vengono caratterizzati sempre negativamente nella narrazione. Parlando di questo, pensando all'intervento che avrei dovuto fare in Aula oggi in dichiarazione di voto, mi sono venute in mente "Le città invisibili" di Calvino, un libro che, come sapete, è stato pubblicato nel 1972, dove l'autore immagina di descrivere delle città e parla di una caratteristica Sicuramente la città di Trude è quella che racconta le periferie, cioè questi contesti urbani sempre uguali a sé stessi. Mi piace leggere proprio le parole di Calvino, perché raccontano cosa sono le periferie nella nostra percezione: «Se toccando terra a Trude non avessi letto il nome della città scritto a grandi lettere, avrei creduto d'essere arrivato allo stesso aeroporto da cui ero partito. I sobborghi che mi fecero attraversare non erano diversi da quegli altri, con le stesse case gialline e verdoline. Seguendo le stesse frecce si girava le stesse aiole delle stesse piazze. Le vie del centro mettevano in mostra mercanzie imballaggi insegne che non cambiavano in nulla. Era la prima volta che venivo a Trude, ma conoscevo già l'albergo in cui mi capitò di scendere; avevo già sentito e detto i miei dialoghi con compratori e venditori di ferraglia; altre giornate uguali a quella erano finite guardando attraverso gli stessi bicchieri gli stessi ombelichi che ondeggiavano. Perché venire a Trude? mi chiedevo. E già volevo ripartire. - Puoi riprendere il volo quando vuoi, - mi dissero, - ma arriverai a un'altra Trude, uguale punto per punto, il mondo è ricoperto da un'unica Trude che non comincia e non finisce, cambia solo il nome all'aeroporto». Ecco,

o per tragedie, come quella accaduta alle Vele di Scampia appena due mesi fa, con il crollo di un ballatoio che ha comportato la morte delle persone che vivevano in quel palazzo, nascono da progettazioni che volevano essere virtuose, da insediamenti urbani che volevano essere architettonicamente e anche dal punto di vista urbanistico, avveniristici. Volevano essere insediamenti urbani che dovevano dare un'impressione di città evolute e moderne. Dove hanno sbagliato all'epoca tanto i sociologi quanto gli urbanisti quanto i governanti nel consentire insediamenti urbani che non avevano collegamenti, che non avevano nulla che consentisse la socializzazione degli abitanti? Con il tempo questi quartieri si sono trasformati in città dormitorio, in città di degrado e di isolamento, dove la carenza, anche dal punto di vista del lavoro, e le difficoltà economiche hanno reso i loro stessi abitanti prigionieri. Non tenere conto di questo e parlare semplicemente di Giornata nazionale per celebrare le periferie urbane, significa fare l'ennesima giornata autocelebrativa, uno *spot*, qualcosa che in sostanza non cambierà in nulla le capacità e le possibilità delle persone che vivono nelle periferie, che pure nel tempo hanno dato prova e dimostrazione di grande volontà di riscatto, con interventi importanti, spesso ad opera delle università italiane, che hanno scelto di delocalizzare in alcuni quartieri delle periferie più degradate - penso a Napoli, ma è successo anche a Roma e in altre città degli uffici, parti delle loro strutture o addirittura facoltà, proprio per consentire in queste città di avere finalmente una vitalità e un senso dello Stato e delle istituzioni che mancavano. Vengo agli ultimi giorni e racconto quello che è stato fatto dal Governo Conte e, ancora prima, dal Governo Renzi, che aveva previsto espressamente un bando per la presentazione di progetti per le periferie urbane, dotandolo di 2 miliardi e 100 milioni stanziati dallo Stato che, con ulteriori finanziamenti, erano arrivati a 4 miliardi. Questo bando, che aveva visto coinvolte le città

e dei sindaci che già avevano ricevuto il finanziamento dei progetti se poi questo bando è stato in qualche modo recuperato, anche se - va detta la verità - non interamente. Dal 2019 bisogna aspettare il PNRR per avere nuovamente un intervento qualificante sulle periferie con i fondi che sono stati destinati saggiamente, intelligentemente e soprattutto con una visione di programmazione, dal PNRR alla rigenerazione urbana. Anche qui però partiamo bene e arriviamo male, perché dalla dotazione originaria del Fondo per la rigenerazione urbana, sono stati tagliati

che si riteneva fossero di importo troppo esiguo, sui 100.000 euro. Questi progetti si è considerato che non fossero coerenti con la programmazione del PNRR, ma sapete che cosa si è tagliato in verità e più di tutto? Si è tagliata la speranza, quella che tanti amministratori locali avevano riposto nei fondi del PNRR, di avere finalmente le risorse per poter dare una risposta ai cittadini per poter riqualificare le periferie urbane e poter dire che finalmente non c'è più una città di serie A e una città di serie B, ma c'è una città che veramente vuole

con molta serenità positiva vivo questo provvedimento, perché anche l'istituzione di una giornata può rappresentare un'attenzione particolare per una configurazione importantissima del nostro Paese: le periferie.

lo spostamento graduale, dolce, intelligente nell'ottica della configurazione staminale, l'inserimento di cellule positive in territori complicati e questo va fatto come priorità, perché

dall'altra possiamo vedere segni complicati, segni regressivi, segni di malattia sociale, nel caso di abbandono, di trascuratezza, di non riconoscimento di un'entità che invece fa parte del territorio in maniera sostanziale. Fa

Come vedete evito il termine "degradati", perché anche l'utilizzo sbagliato del lessico può marcare a fuoco un territorio; parlo di territori complicati, di territori complessi, ai quali dobbiamo veramente

ma anche come chi ha presentato il provvedimento, che le *chance* per invertire la rotta esistano e siano anche molto forti, ma certo bisognerà agire in maniera economica

degradante e regressiva. Evitiamo polemiche, per una mobilitazione che ci deve vedere tutti, in queste realtà, dare alla periferia

la relatrice che ha ispirato il provvedimento, ci mancherebbe. Anzi, magari proprio le periferie meriterebbero qualche elemento di approfondimento, però dico onestamente che non esprimeremo mai più voto favorevole a qualunque Giornata

Bisognerà inventarsi le mattinate, i pomeriggi, le sere.

su argomenti molto significativi. Per esempio, arriveranno la Giornata nazionale del panettone italiano, la Giornata nazionale della cultura motociclistica, la Giornata nazionale del riciclo della carta, la Giornata nazionale dei figli d'Italia

Perché in Italia è diventata straordinariamente importante la Giornata della memoria, tanto per dirne una? *(Applausi)*. Tutti sappiamo che si celebra il 27 gennaio e intorno a essa è stata costruita negli anni una straordinaria narrazione. Come ho detto spesso in quest'Aula,

perché si discute di un grande fatto storico straordinario intorno al quale bisogna giustamente costruire le coscienze. Non vi viene il dubbio che istituire,

come le Giornate, così come sono state concepite negli anni passati, si fa un danno enorme alle nuove Giornate che saranno istituite (e che io non voterò più, come vi ho annunciato), ma soprattutto a quelle che già esistono e che sono veri momenti formativi per le coscienze del Paese. Francamente a me questa pare una cosa

Signor, Presidente, pur condividendo quello che ha appena detto il collega De Cristofaro, anche sul numero delle delle giornate che sono state istituite e che sono in fase di istituzione, credo che questa di oggi sia però nel merito una di quelle giornate che è utile approfondire come argomento, perché tocca il cuore delle nostre città e ancora di più delle persone che vivono nelle periferie. Milioni di italiani, circa il 35 per cento della nostra popolazione e anche più, vive nelle periferie. Se consideriamo oggi il concetto di globalizzazione, la periferia ha subito un'ulteriore trasformazione. Infatti le periferie non sono più solo le aree marginali delle città, ma spesso si trovano nelle zone rurali, si trovano nelle aree che non sono interconnesse con le grandi reti immateriali, dove i cittadini non hanno accesso ai servizi. Parlavamo poco fa delle zone montane, che spesso sono, per i piccoli borghi almeno, oggetto di spopolamento, di tutti quei posti, insomma, dove non c'è accesso non solo ai servizi ma anche alla cultura, ai grossi centri culturali. Non ci sono siti dove si fa istruzione di qualità. Molte persone, molti cittadini oggi vivono in questi contesti, quindi non è solo un fatto geografico ma un fenomeno sociale. Queste aree non sono solo case, ma sono luoghi che si intrecciano con la difficoltà della vita quotidiana e con la forza delle comunità. Sono le contraddizioni della vita delle persone che vivono nelle città e ancora di più nelle periferie, che spesso sono dipinte come luoghi di degrado - lo abbiamo visto anche negli interventi precedenti - abbandonati dallo Stato, con le persone che vivono ai margini, lontane dai centri decisionali, dove si decide il futuro del nostro Paese. Dietro questa immagine stereotipata, però, c'è una realtà più complessa in molti casi anche straordinaria. Le periferie non sono solo spazi di marginalità, ma sono anche spazi di resistenza e di creatività. Sono nate, lo sappiamo, quando le nostre città esplodevano, dopo l'industrializzazione. Sono state zone cuscinetto fra i centri e le zone rurali. Molte di queste aree sono state costruite senza piani, alcune sono state costruite con piani inadeguati, inadeguati, che rispondevano all'ideologia della casa collettiva, quindi quartieri periferici senza identità, senza riconoscibilità, con questi fabbricati che adesso in alcuni casi si chiamano lotti come se i cittadini dovessero vivere in contesti che hanno dimostrato di essere di degrado, dove c'è insicurezza sociale e insicurezza urbana.

possono diventare anche molto di più rispetto a quello che noi pensiamo. Possono entrare forse anche un motore di rinascita culturale e sociale del nostro Paese. Dove mancano le infrastrutture e anche le risorse forse fioriscono, anzi spesso fioriscono forme di solidarietà e di creatività che al centro forse non si possono neanche immaginare. Pensiamo alla musica *rap*, che è nata nei sobborghi di New York, alla *street art*, al cinema, al neorealismo italiano, ai film di De Sica e di Rossellini, alle opere di Pasolini, che riguardano quei contesti dove c'era, sì, violenza e privazione, ma anche una cultura autentica non ancora corrotta dalla modernità, resiste a questi spazi più consumistici. Sono spazi di resistenza culturale, dove sopravvivono le tradizioni popolari, dove quindi si può scoprire spesso un'umanità molto più pura, molto più viva. Dalle periferie può dunque

dove si possa costruire un futuro basato non solo sulla coesione sociale, ma anche sulla creatività e sulla sostenibilità. Ci sono molti esempi europei, a partire da Friburgo, che è diventata la capitale europea delle città che hanno attuato i principi di rigenerazione urbana all'interno di aree che erano marginali, sperimentando attività che oggi sono riproposte anche in Italia: gli orti urbani, i percorsi ciclabili, gli spazi condivisi. Nelle periferie nascono nuove sfide di rigenerazione urbana integrata, puntando anche sulla cultura e sull'istruzione - come dicevo prima - e favorendo l'accesso alla cultura con centri culturali, biblioteche, teatri, scuole di alta qualità. Dobbiamo partire dagli esempi presenti in Europa, in cui ci sono già non solo gli eco-quartieri, ma addirittura le eco-città. Citavo prima Friburgo, ma c'è anche il caso di Bilbao, dove con un museo si è rigenerato un intero quartiere, puntando alle infrastrutture di mobilità e agli altri servizi culturali. Da sindaco, intrapresi azioni che riguardavano la

Spero che questo sia solo un momento, perché è un dibattito molto trascurato nel nostro Paese, mentre negli altri Paesi europei è molto più avanti, come dicevo prima. Credo quindi che questo disegno di legge, promosso dal collega Battilocchio, rappresenti almeno un primo passo rispetto a questa tematica. Proponendo la Giornata nazionale delle periferie urbane si può offrire alle istituzioni e ai cittadini un'occasione concreta per concentrarsi sul tema

del futuro deve partire dai margini per coinvolgere tutti. Questo può essere un buon punto di partenza per una vera rinascita. Per questi motivi dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo all'istituzione della Giornata nazionale.

comincia a diventare un po' pesante la continua istituzione di giornate nazionali. Mi viene in mente un detto popolare: il dire è nemico del fare. Qui continuiamo a proclamare giornate, salvo poi, oggettivamente, non fare nulla nella direzione di risolvere quelle che, evidentemente, sono delle criticità. Comunque, il concetto di periferia si individua in contrapposizione a quello di centro. Entrambi fanno parte del medesimo organismo. Quindi possiamo pensare, come in questo caso, alle periferie urbane come come organismo della città, ma anche alle periferie sociali, a quelle economiche e a quelle culturali, che spesso coincidono. Io parlo per esperienza diretta. Io sono nata, cresciuta e tuttora vivo nella periferia di una grande città come Milano e ne conosco benissimo le problematiche. Se la periferia è periferia rispetto al centro patinato della città, capita che le periferie diventino, viceversa, il centro di un altro organismo, di altri organismi, che sono quelli della delinquenza, della criminalità, del disagio sociale e della povertà. povertà. In una città come Milano, alle ore 20 scatta la tolleranza. Compaiono, in tutte le vie della città, sia quelle centrali che quelle periferiche, tende, sacchi a pelo e i disagiati, i senzatetto, i poveri si organizzano per trascorrere la notte. Mi è capitato a largo Corsia dei Servi, in pieno centro di Milano, di vedere una coppia - potevano essere i miei vicini di casa un *trolley* dell'aeroporto si sistemavano con i sacchi a pelo per passare la notte. È chiaro che questa periferia sociale non può più essere trascurata. Se noi non curiamo anche gli aspetti periferici di un organismo, l'intero organismo, dopo un po' di tempo, ne risentirà. Infatti, tutti i fenomeni di delinquenza, che coinvolgono tutti i cittadini, hanno anche questa derivazione. Ma cosa sono le periferie urbane? In pratica, sono contesti situati ai limiti della città, molto vicine alle arterie principali di comunicazione, che risentono di un forte inquinamento, sia acustico sia atmosferico. Sono caratterizzate da costruzioni del *boom* economico degli anni 60 e 70; quindi, edifici economici che, visto il trascorrere del tempo, avrebbero sicuramente bisogno di una rigenerazione. Non ci sono più centri di aggregazione sociale, perché, nelle

Purtroppo, con la speculazione edilizia, le aree rurali sono state aggredite dalla cementificazione, e spesso sono stati costruiti grandi centri commerciali, piuttosto che centri

invece che su politiche del celebrare. Quindi, se abbiamo problemi di senzatetto, significa che non ci sono sufficienti case popolari, che non c'è l'*housing* sociale e che bisognerebbe investire nella casa per i poveri. Manca totalmente il verde e i nostri anziani sono praticamente sigillati in un blocco di cemento; non ci sono spazi verdi per avere il contatto con la natura; i fondi per la riforestazione urbana del PNRR sono stati tagliati, tagliati, perché i Comuni dicono che non hanno sufficienti spazi dove piantumare gli alberi. Se andiamo però a vedere i piani regolatori di quei Comuni, scopriamo che nelle aree identificate e destinate all'edificazione in realtà ci sono suoli liberi, naturalmente rinaturalizzati e che, anziché essere destinati alla nuova cementificazione, dovrebbero costituire quei polmoni verdi per la città di cui tutti potrebbero usufruire e beneficiare, compreso chi vive nei quartieri periferici

grave. Non ci sono misure e investimenti sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Chi vive nei quartieri periferici e semiperiferici è praticamente soffocato dall'inquinamento trecento giorni l'anno, e non ci sono politiche per ridurre le emissioni. Ad esempio, banalmente il riscaldamento degli edifici è quello che comporta il maggior incremento dell'inquinamento. Si è tolto il superbonus, ma non si è fatto nulla in questa direzione. Quindi siamo - ahimè - in una situazione gravissima. Sto seguendo il disegno di legge sulla rigenerazione urbana, e noi del MoVimento 5 Stelle ne abbiamo presentato uno, ma onestamente nel testo del relatore non si vede nulla che vada in tale direzione; nulla che pensi alla rigenerazione urbana anche dal punto di vista sociale. Si danno incrementi volumetrici a iosa, non si pensa a tutelare gli aspetti sociali e ambientali, e io spero di riuscire a fare una discussione produttiva e proficua con il relatore, per cercare di portare a casa quantomeno una rigenerazione urbana che consideri aspetti importanti della società. Mi rivolgo quindi al Governo: occorre fare. Basta parole: bisogna agire.

non possa che dimostrare anche a chi ci sta seguendo da casa l'attenzione di questo Governo per le specificità del nostro territorio, che è veramente molto veramente molto vario anche nelle sue problematiche. Passiamo da un problema relativo alle zone di montagna, ossia lo spopolamento, al sovraffollamento di cui soffrono tante nostre periferie. E quando parlo di periferie, non mi riferisco

Devo però anche dire - come abbiamo poi ricordato in 1a Commissione - che questa è una Giornata che ha un significato un po' differente, perché il testo è stato fortemente voluto da tutti i

alla Camera, per dare vita alla Giornata, con il lavoro che sta dietro a tutto questo e, quindi, il grande lavoro che sta facendo la Commissione. Ma non è tutto. Sempre per dimostrare che l'istituzione di questa Giornata proprio con un nostro emendamento a firma Lega abbiamo chiesto e ottenuto dal Governo, soprattutto grazie alla disponibilità del Ministero dell'interno, la creazione dell'Osservatorio sulle periferie. Vi devo dire che l'idea di proporre l'emendamento, che poi è stato approvato, è nata proprio dal fatto che al decreto Caivano veniva contestata un'attenzione forse eccessiva per alcune zone - ovviamente che aveva urgente bisogno di un intervento - e poca attenzione per altre zone del Paese che hanno problematiche simili o che comunque, in una graduazione di problemi, possono avvicinarsi a Caivano.

di partecipanti. Si occupa della promozione di iniziative volte all'analisi e alla riqualificazione delle zone degradate, di interventi di formazione alla cultura della legalità (con un occhio di riguardo per le fasce giovanili), incentivare lo scambio di informazioni fra i diversi attori e di fornire supporto ai soggetti sia pubblici che privati. Questo Osservatorio si sta già organizzando per lavorare al meglio,

è stato rispettato l'impegno del Governo e del Ministero dell'interno: l'Osservatorio c'è e sta iniziando a lavorare. Cosa abbiamo fatto, sempre nell'ottica di dare concretezza a questo provvedimento, periferie urbane il 24 giugno di ogni anno? In occasione dei lavori della Commissione, come Gruppo Lega abbiamo presentato un ordine del giorno, che è stato accolto come raccomandazione dal Governo, volto a creare un collegamento tra il lavoro dell'Osservatorio e la Giornata delle periferie. L'Osservatorio ha fra i suoi compiti rendere una relazione annuale sui risultati ottenuti. E abbiamo chiesto al Governo di coinvolgere l'Osservatorio nell'organizzazione della Giornata delle periferie, anche rendendo noti i risultati di ogni anno e poi per collaborare a varie iniziative. Credo che questo dimostri veramente una grande attenzione sul problema delle periferie. Come dicevo prima, siamo passati dalla montagna alle periferie, con problemi completamente diversi, ma ricordiamoci che nessuno di noi sceglie dove nascere

ci ha illustrato le bellezze della montagna e la fortuna di vivere in montagna. Chi vive in una periferia degradata non ha scelto di nascere e di vivere lì

innocenti ovviamente, di scelte poco lungimiranti - per usare un eufemismo - che sono state fatte soprattutto negli anni del *boom* economico, quando c'era bisogno di trovare un posto per tante famiglie che necessitavano urgentemente di un alloggio, senza pensare però a dotare quelle zone di servizi. E poi sappiamo tutti quello che è successo e come siamo arrivati ad oggi. Non solo dobbiamo evitare che la situazione peggiori, ma dobbiamo cercare - così ha già cercato di fare questo Governo, ma anche i Governi precedenti - di dare delle risposte e di mettere in atto delle iniziative che vanno dalla sicurezza alla alla riqualificazione urbana. Ricordava la collega tutto quello che è stato fatto e che è ancora in atto con il PNRR, ma ci sono sicuramente tante altre cose che possono essere sviluppate, con un'attenzione ai singoli territori, perché le periferie non hanno tutte gli stessi problemi. Gli interventi che devono essere fatti nelle zone periferiche o nei quartieri degradati, anche se non così periferici, delle nostre città non sono gli stessi. Credo che l'attenzione sia dimostrata da tutta la serie di provvedimenti che sono stati portati avanti da questo Governo, anche con la collaborazione delle opposizioni, che è fondamentale. Ricordiamo sempre che il lavoro più importante e più umanamente impattante è quello che viene fatto sui singoli territori, non solo dalle istituzioni che sono importanti - un occhio di riguardo va sempre dedicato ai nostri Comuni, che hanno bisogno sicuramente di essere valorizzati e aiutati, soprattutto nei contesti più difficili - ma anche dal terzo settore, dalla scuola, dalle parrocchie e dalle associazioni, che danno un

a prevalenza agricola, con tanto verde, dove i bambini possono uscire a giocare senza grandi pericoli, ci sono però delle cose belle da valorizzare anche nelle nostre città e nelle loro periferie, persino in quelle che vivono un maggior degrado. Abbiamo degli esempi - come abbiamo visto quando abbiamo fatto le audizioni del decreto Caivano - dell'impegno che viene messo sui territori rischiando la propria vita. È triste ascoltare in audizione chi ti racconta che, per arrivare a scuola, deve attraversare diverse piazze dello spaccio. Non è un problema che c'è solo Caivano. Purtroppo il problema c'è, ma ci sono anche tante persone che donano la loro vita e il loro tempo per aiutare i loro concittadini, i nostri bambini. Per questo motivo dichiaro il voto favorevole da parte del Gruppo Lega

Signor Presidente, ci troviamo oggi ad affrontare un tema di enorme serietà, che però sta dentro un contenitore che di serietà ne mette fuori e ne esprime veramente poca. Io potrei fermarmi o ripetere le cose che ho sentito dal collega De Cristofaro per argomentare la ragione per cui il Gruppo Partito Democratico si asterrà su questa proposta di legge. di legge. Non scendiamo in battute, leggendo a voce alta l'elenco delle giornate: mi limito soltanto a quella della ecospiritualità, che è in arrivo ed è ancora da assegnare, ma ognuno di voi può andarsi a leggere il lunghissimo elenco di giornate, gran parte delle quali anche molto discutibili per la loro scelta. Penso a quella della

noi poi ha orientamenti e una cultura e, quindi, potrebbe anche essere che non tutti siamo in grado di apprezzare le proposte di altri

Quest'ultima è un po' come gli amici: non si può essere amici di tutti, come mi dicevano da bambina, perché finisce che non sei più amico di nessuno. Ecco, noi abbiamo ormai più giornate da celebrare che giorni nel calendario e questo finisce con lo svilire enormemente il tema che quella giornata propone. Intanto perché passa inosservata. Io vi sfido a provare a chiedere a chiunque se sa quali sono le giornate che si celebrano nel nostro Paese, a parte quelle davvero molto importanti. Nel caso specifico, questo è davvero un peccato, perché quello delle periferie è un tema di primaria importanza. La rigenerazione delle periferie è davvero la sfida che il Paese deve affrontare tra le tante, ma certamente è una di quelle che va in testa. Quelle periferie, che ormai qualcuno ha anche definito periferie dell'anima, sono il luogo in cui noi siamo chiamati a misurarci con una molteplicità enorme di problemi drammatici che vanno dalla disuguaglianza alla povertà, dalla dispersione scolastica al degrado e alla violenza. C'è di tutto ed è sotto i nostri occhi continuamente. Ed è per questo che questo tema merita e meritava di essere affrontato.

risorsa un programma di intervento per le periferie, perché alla fine è davvero soltanto un'operazione propagandistica che ripropone, quindi, una celebrazione vuota. Questa celebrazione è stata fissata al 24 giugno. Io sono davvero curiosa di andare a vedere il prossimo 24 giugno che cosa succederà. Ma quello che non succederà è che venga affrontata, appunto, la sfida delle sfide. Come è stato richiamato poco fa dalla collega, invece, invece, a conferma di quello che dicevo, stiamo davvero affrontando un tema importantissimo, che è la rigenerazione non solo di uno spazio geografico, ma anche di un tessuto sociale prima di ogni altra cosa a seguito di questa azione di rigenerazione, partirà poi anche la rigenerazione geografica dei luoghi e delle sedi. Siccome, tra l'altro, abbiamo istituito - in maniera secondo me molto intelligente e saggia - la Commissione parlamentare sulle periferie,

collegato a una significativa nuova edizione di politiche abitative, anche con il rilancio della locazione - resta uno dei temi che ci interroga, penso, anche individualmente tutti i giorni, perché credo che chiunque di noi conosca persone che si devono confrontare con il dramma di trovare una casa e di trovare una casa dignitosa - e con un rinnovato sforzo per qualificare le politiche sociali

sociale. Molto importanti sono le proposte che via via nel tempo sono state fatte nel nostro Paese proprio sul tema delle periferie. Voglio ricordarne, tra le altre, una che è di Fabrizio Barca, che nella sua Urban@it ha suggerito di formare giovani agenti di sviluppo da impiegare in 200 quartieri delle città italiane dove più grave è il disagio.

un comitato di sorveglianza in cui coinvolgere le Città metropolitane e una mappa delle aree di intervento. Ma voglio anche ricordare che, tra le proposte serie, serie, molte si sono trasformate in esperienze importanti che si vanno moltiplicando, per fortuna anche con il sostegno delle università che, da sole o con associazioni e fondazioni, hanno cominciato a riflettere e quindi a offrire davvero al legislatore una grande quantità di strumenti, di idee, di possibili iniziative che invece questa Giornata finisce poi con il liquidare senza una risposta, come investire in questioni ambientali e sociali (queste due cose si incrociano spesso); riutilizzare spazi abbandonati per attività culturali; promuovere nuovi lavori; la rimessa in produzione di terreni agricoli; la formazione di comunità energetiche; forme imprenditoriali come le cooperative di comunità. Voglio qui ricordare che

coloro che vivono in quelle periferie, dove nulla è cambiato e dove nulla sta cambiando e che - ammesso che ne siano informati, ma so che il disegno di legge propone anche una Giornata di informazione

ci sono esperienze importantissime anche in paesi del Nord che ci hanno insegnato che dove ci sono la periferia e il degrado sociale

ma al tempo stesso non ci sentiamo di poter condividere la scelta di liquidare un tema così importante con l'istituzione dell'ennesima Giornata. Anche noi ci associamo alla preghiera di chi dice: per favore, prima di continuare a istituire una Giornata dopo l'altra, proviamo a fare qualcosa di concreto.

Noi pensiamo - e annuncio fin d'ora il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia a questo provvedimento - che provvedimenti come questo possano essere utili se, come in questo caso, fanno parte di un percorso.

hanno sottoscritto questo provvedimento. *(Applausi)*. Se alla Camera lo sottoscrivete, non potete poi venire al Senato a dire che è un provvedimento inutile, se non addirittura dannoso. Tutti però sono stati concordi nel dire che il tema trattato è assolutamente importante. Ricordo che questa Giornata viene fissata

sociale è importante e complesso. È un tema che si affronta con un approccio multidimensionale, sicuramente intervenendo dal punto di vista materiale, ripensando anche i luoghi fisici, spesso mal pensati, peggio realizzati e peggio ancora manutenuti, ma anche lavorando sul valore e l'impatto immateriale delle trasformazioni urbane e sociali, che sono necessarie per rigenerare realmente le periferie, per cambiare i luoghi, per trasformare luoghi privi di punti di riferimento e di senso di appartenenza ad una comunità in luoghi dove invece ci sia qualità della vita. Da questo punto di vista, a coloro che hanno detto che si declama solo la giornata - in questa legislatura, il Governo Meloni e questa maggioranza hanno avviato un percorso importante da questo punto di vista. C'è un esempio molto preciso che si chiama esempio Caivano. esempio Caivano. Ho ricordato solo una delle tragiche vicende che hanno riguardato quella comunità, dove non c'era assolutamente la presenza delle istituzioni, dove non c'era senso di appartenenza, dove c'era degrado assoluto, lo Stato è tornato, ha fatto sentire la sua presenza. *(Applausi)*. Ha messo insieme le comunità locali, le istituzioni, le parrocchie, le associazioni sportive, il volontariato sociale, le imprese e ha messo in campo un'azione, un approccio integrato che è l'unico modo per restituire qualità della vita e dignità alle periferie urbane. Allora, oggi, dove c'era il degrado più totale, a Caivano, la speranza divampa. Questo modello può essere replicato, ovviamente con il dovuto adattamento alla specificità e alle identità locali, e sarà replicato. Il modello Caivano sarà replicato in tante e tante periferie altrettanto problematiche. Si fonda sul tema della consapevolezza dell'appartenenza e della consapevolezza civica, della capacità di coinvolgere i cittadini, di farli sentire parte di qualcosa. Vedete colleghi, un giardino curato non è solo un esempio magari di buona amministrazione, di buona manutenzione: è un segnale per un cittadino che abita in quel quartiere, è un segnale di speranza per il futuro. Le periferie urbane, come intese nell'epoca moderna, sono fondamentalmente la negazione stessa del concetto di città. Quindi, la periferia in questo senso parte sconfitta in partenza, perché nega in radice la possibilità di appartenere a qualcosa, di sentirsi parte di una comunità. Abbiamo tanti, tantissimi esempi, esempi, partendo dalla Capitale, che ovviamente è la mia appartenenza territoriale. Tutti conoscono la realtà di Tor Bella Monaca, tutti conoscono il cosiddetto serpentone di Corviale, ma ci sono nella Capitale e in tutta Italia tanti e tanti altri esempi, magari meno noti, di quartieri figli spesso anche di una impostazione

all'architettura e al vivere comune del marxismo. Tra questi tanti quartieri, ce n'è uno che, pensando a questa dichiarazione di voto, mi ha ricordato un film un film che tutti conoscono, «Caro Diario» di Nanni Moretti, nel quale a un certo punto, nel suo peregrinare in motorino, Nanni Moretti si ferma in un quartiere, situato a Roma Sud - Spinaceto - e dice: Spinaceto, me lo aspettavo peggio. Il problema è che poi Nanni Moretti prende il motorino e se ne torna in altri lidi. I cittadini di Spinaceto, delle mille Spinaceto di tutta Italia rimangono lì, con quei progetti fallimentari, con quelle manutenzioni che non ci sono mai state, con quelle promesse che non si sono mantenute. Quindi la periferia o diventa comunità cittadina oppure resta un non luogo, nel quale è impossibile sentirsi a casa propria. E, se non ci si sente bene a casa propria, è anche difficile immaginare di fare qualcosa di bello della propria vita. È proprio per questo che noi dobbiamo agire con forza su quegli agglomerati senza anima che sono un po' spazi in tutta Italia: a Napoli con Scampia, con Scampia, e Palermo con Zen 2, a Modena con il complesso R-Nord, a Cagliari con Sant'Elia, a Genova con la Diga di Begato sulla quale però si sta facendo, grazie al centrodestra, un'importante opera di rigenerazione, a Bari con il quartiere San Paolo e potrei continuare all'infinito. C'è un architetto paesaggista, Leon Krier, che definisce molto bene cosa possono essere queste periferie: «La città disegna sempre i suoi limiti, definisce lo spazio urbano da quello rurale. La periferia, invece, non disegna nulla, dichiara che tutto può essere di sua pertinenza. La periferia odia se stessa, sa di essere né campagna, né città, non riesce quindi a vivere in pace con se stessa». Ecco, noi dobbiamo lavorare su questo. Colleghi, alcuni di voi hanno citato il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Vi segnalo che è grazie a questo Governo che sta andando avanti, con grandi risultati anche se, alcuni Comuni governati dalla sinistra hanno perso, in quell'occasione, la grande opportunità di attuare una rigenerazione urbana e in alcuni casi hanno pensato, come a Roma, Giunta Raggi, scelta poi confermata dalla Giunta Gualtieri, di utilizzare quei progetti per dare la casa in modo ufficiale a chi l'aveva occupata. Questa non è rigenerazione urbana, questo non è quello che immaginiamo noi.

un po' abusata - "rigenerazione urbana" nel senso di farla passare dalla poesia alla prosa, iniziando a dare strumenti concreti alle Regioni e agli enti locali per realizzare questi progetti di rigenerazione, che in alcuni casi però - e questo è importante necessitano di essere non di mera rigenerazione; infatti, quando una cosa è progettata male o in modo sbagliato, esiste la soluzione della sostituzione edilizia: demolire e ricostruire.

ma ci dobbiamo lavorare e lo stiamo facendo. È quello di riportare equilibrio in questa contraddizione irrisolta da decenni nelle grandi periferie urbane. È una grande sfida, ma con un approccio integrato e con la continuità dell'azione, ripartendo, come ho detto, dall'esempio di Caivano, esportandolo in tante altre situazioni e adattandolo, possiamo riuscire a curare e risanare, sia esteriormente, sia interiormente, le periferie della nostra Italia e restituire loro un'anima e un senso di appartenenza alla comunità nazionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, farò una breve introduzione, cercando di illustrare la relazione che, come è stato detto, è in distribuzione un momento importante dal punto di vista del lavoro svolto dalla Commissione che ho l'onore di presiedere. Arriviamo a questa relazione all'Assemblea in modo unitario: vorrei infatti sottolineare che la

il dato fondamentale è che ognuno di loro, giustamente, risponde ai propri dirigenti e alle proprie indicazioni, ma non c'è una *governance* unitaria:

per intervenire, ma, nello stesso tempo, ognuno lavora in modo verticale e risponde giustamente alla propria indicazione. Il dato vero che emerge è sostanzialmente il fatto che

o allo stesso Giubileo a Roma: c'è un accordo tra le istituzioni locali e tutti i soggetti abilitati a intervenire in questa direzione e le parti sociali svolgono un ruolo fondamentale. ruolo fondamentale. Visto e considerato che anche in Regione Lombardia c'è una Commissione d'inchiesta e che il Comune di Milano ha dimostrato un interesse in questa direzione, abbiamo pensato e stiamo lavorando

La vicenda pandemica ci ha posto di fronte al fatto che molte realtà (le fabbriche) all'inizio si dovevano chiudere, per la situazione che c'era; invece una concertazione tra le parti ha portato ad affrontare i temi i temi e a dare una risposta positiva in questa direzione. Quando si dice che bisogna alzare il livello della cultura della sicurezza, è necessario fare in modo che i soggetti territoriali che sono preposti a queste funzioni abbiano

Se è possibile fare un protocollo di fronte alle grandi opere, perché non farlo anche sul cantiere diffuso? La domanda è questa. È molto più difficile il cantiere diffuso su una Provincia, però bisogna provarci e fare in modo che si vada in questa direzione,

Questo è in contrasto con la questione degli appalti e dei subappalti. Molti degli incidenti che sono successi e succedono sono determinati dagli appalti e dai subappalti,

Avverto che eventuali proposte di risoluzione al documento in esame potranno essere presentate entro la conclusione della discussione. Dichiaro aperta la discussione. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. non si può morire per lavoro, non si può uscire di casa e non ritornare più nel 2024. Ce lo siamo già detti, l'abbiamo detto dopo l'incidente di Brandizzo, dopo l'approvazione della mozione all'unanimità in quest'Aula, dopo i vari incidenti (ne succedono quasi tre, purtroppo, ogni giorno), dopo quello di Firenze e dopo quello di cui parlerò ancora nel corso del *question time*, ovvero l'incidente alla Toyota dell'altro giorno. Non sono numeri, come ha detto il presidente Magni: non dobbiamo parlare di numeri, né di statistiche, ma dobbiamo ricordarci che dietro questi incidenti ci sono donne e uomini e ci sono figli, ci sono figli, anche non ancora nati, che non vedranno mai il loro padre o la loro madre. Sono tragedie che colpiscono famiglie. Noi dobbiamo essere responsabili su questo. Ecco perché la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni del lavoro, di cui faccio parte, con molto senso di responsabilità ha lavorato unitamente (e per questo ringrazio i colleghi, il presidente Magni e il vice presidente Dreosto), considerato che la questione non è deferibile e necessita di essere affrontata non solo mediante l'introduzione di ulteriori interventi normativi, ma soprattutto attraverso misure pratiche ed effettive in grado di incidere sull'operatività del sistema della sicurezza sul lavoro. L'analisi della Commissione ha evidenziato che l'esternalizzazione dei lavori e dei servizi in appalti o subappalti è pericolosa, perché permette di ridurre al minimo la responsabilità che viene distribuita su una miriade di soggetti che rendono sempre più difficile la comunicazione interna e allo stesso tempo i ritmi sono insostenibili, evidenziando sempre più la fragilità dei contratti dei lavoratori. lavoratori. Un altro problema è quello della molteplicità delle forme di lavoro irregolare, soprattutto i contratti pirata o quelli che vengono applicati, sebbene la mansione che la persona viene chiamata a svolgere non sia quella coperta dal contratto stesso. Ci vuole quindi responsabilità responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti: il committente privato, l'appaltatore, i subappaltatori e i lavoratori. Spesso gli incidenti non derivano da una carenza formativa o informativa, ma sono una conseguenza di lacune progettuali, di mancanza di coordinamento delle lavorazioni o di tempistiche incompatibili con la natura e la complessità degli interventi. Occorre quindi una *governance* negli appalti sia privati sia pubblici. Ecco perché solo attraverso l'utilizzo di organizzate procedure si garantiscono efficienza ed efficacia del sistema e come Commissione monocamerale sulla sicurezza del lavoro abbiamo anche portato avanti un'analisi attenta e oltre alla *governance* è stato ribadito che la condotta umana non risulta mai la causa esclusiva o principale dell'infortunio. Per questo serve una cultura della sicurezza sul lavoro

un progetto di studio e intervento per migliorare le condizioni di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Il progetto di studio si sviluppa in una duplice direzione: da un lato, c'è il tema della *governance* dei sistemi complessi e, dall'altro, quello della diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, coinvolgendo però anche tutti i soggetti che entrano a diverso titolo nel complesso sistema del lavoro, della prevenzione e della sicurezza. Ecco perché la Commissione ha voluto direttamente al tavolo e ha iniziato a lavorare con la commissione sicurezza sul lavoro della Regione Lombardia e del Comune di Milano, e del Comune di Milano, che sono già organizzate, per sperimentare come approccio condiviso un paradigma della sicurezza, sperimentandolo direttamente in quest'area geografica, facendo in modo che poi si possano delineare linee guida quali *best practice* che possono essere utilizzate in altre realtà. Verranno analizzati anche i sistemi complessi e positivi nei diversi settori per portarli all'attenzione nell'elaborazione di queste linee guida. Il tutto verrà realizzato tramite la sperimentazione, che può apportare modifiche anche all'organizzazione, nel momento in cui si inseriscono anche innovazioni tecnologiche. Per questo è stato considerato anche l'uso dell'intelligenza artificiale all'interno dei sistemi lavorativi. La sperimentazione in situazioni nuove e diverse, in contesti e settori diversi servirà anche a valutare l'opportunità di potenziare l'attività di controllo per le condizioni di lavoro dei prestatori di opera attivi in base a regimi contrattuali di appalto e subappalto. però importante incentivare la disseminazione, cioè quella parte di divulgazione e diffusione che deve essere fatta a tutti i livelli. Vi porteremo direttamente in Aula questa esperienza per poterla condividere tra noi colleghi a livello di tutte le istituzioni, con i Ministeri. Ritengo importante la diffusione di queste linee guida all'interno

tra le due Commissioni. Infatti, fare eventi per tre giorni parlando di sicurezza sul lavoro, con la partecipazione direttamente del presidente Mattarella in un solo ramo del Parlamento, è molto bello e fa *audience*, ma non porta azioni concrete e reali per la vera sicurezza dei lavoratori. poche parole, ma fatti concreti e sono contenta dell'avvio di questo progetto sperimentale per la tutela di tutti i lavoratori, perché non si può morire di lavoro nel 2024.

questo percorso. È già stato raccontato il metodo con cui la Commissione ha lavorato. Abbiamo svolto audizioni e doverose analisi di dati, statistiche e relazioni degli enti preposti, nonché fatto diverse missioni dal Nord al Sud del Paese. Avremmo potuto limitarci a indicare come risultanti del lavoro svolto alcune criticità, che pure non non mi esimerò dal menzionare e indicare, ma la Commissione ha voluto fare un passo in più. Oltre all'attività di inchiesta, che porta alla denuncia di cause critiche e possibilità di intervento, ha voluto proporre, come è stato già ricordato, un modello sperimentale e ha voluto indicare alcune *best practice.* Non era dovuto e non sempre le Commissioni d'inchiesta arrivano a questo, ma in questo caso penso sia l'originalità di questo lavoro a offrire un contributo non soltanto soltanto al lavoro parlamentare che continuerà, ma anche al Governo (se, come spero, vorrà fare tesoro del percorso che il Parlamento ha fatto in maniera unitaria, cosa

che oggi voteremo, saranno ancora oggetto, spero, di intervento da parte del Governo e del Parlamento. Il primo elemento è quello dei controlli. Sappiamo che, purtroppo, gli organici dell'Ispettorato del lavoro sono sottodimensionati

perché gli stipendi dei dipendenti pubblici, ahimè, non sono competitivi rispetto all'inflazione. Sappiamo anche che la ministra Calderone ha indetto un nuovo concorso per 750 unità che, se avrà

e lo è ancor di più se consideriamo che, quando i controlli vengono fatti, l'efficacia c'è. Pensate che dopo il tragico incidente nelle campagne di Latina, in cui ha perso la vita un lavoratore indiano, Singh, amputato di un braccio e abbandonato, la campagna

Il secondo aspetto, già citato dalla collega Murelli (e mi fa piacere che si converga da partiti politici diversi su questo punto), è quello della criticità della catena degli appalti e dei subappalti. Noi sappiamo da tempo che la frammentazione del ciclo produttivo non è soltanto una ragione di abbassamento delle condizioni salariali e delle condizioni generali dei lavoratori, ma è anche un fattore di criticità per la sicurezza. Non è un caso che i diversi incidenti mortali - ahimè, a volte anche multipli - che abbiamo purtroppo registrato negli ultimi mesi, siano avvenuti in situazioni complesse, dove il ricorso agli appalti e ai subappalti era stato significativo. Ricordiamo che nel tragico caso del cantiere di Firenze si sono contati più di sessanta tra appaltatori e subappaltatori, quindi vi era un elemento di estrema non soltanto per le condizioni di lavoro e per la sicurezza sul lavoro, ma spesso anche per la sicurezza dei cittadini e degli utenti. Voglio citare qui - ma non in termini polemici, perché non è questo il contesto - alcuni gravi incidenti che sono avvenuti sulla rete infrastrutturale ferroviaria in particolare, in cui il coinvolgimento di un gran numero di appaltatori e subappaltatori ha determinato criticità di sicurezza generale anche per i cittadini. Questo è un punto ulteriore che è emerso dalla nostra attività e rispetto al al quale ci siamo sforzati di dare risposte in termini propositivi e costruttivi, indicando delle buone pratiche, che sono state ovviamente già citate dal presidente Magni e che troverete nella relazione finale. Voglio ricordare, anche per ragioni geografiche e di coinvolgimento personale in alcuni di questi percorsi, quando sono stata assessora al lavoro al Comune di Milano, il caso di Expo e di M4, con la rete di sicurezza di protocolli costituiti anche grazie grazie alla collaborazione tra istituzioni e organizzazioni sindacali e dei lavoratori e l'introduzione di strumenti anche di natura digitale. Penso alla banca dati di legalità, la piattaforma di legalità che è stata utilizzata per Expo e per M4, che è stata uno strumento in grado al tempo stesso di contrastare infiltrazioni malavitose nella catena di questi grandi eventi e di garantire un controllo meticoloso delle presenze nei cantieri, della nazionalità dei lavoratori e degli orari di frequenza del cantiere. Strumenti come questi, che peraltro sono previsti anche come obbligatori per gli appaltatori che utilizzano protocolli di legalità, dovrebbero essere più diffusi e noi li abbiamo citati come buone pratiche. La questione della *governance* di situazioni complesse credo sia il punto d'arrivo più significativo del percorso che abbiamo fatto, cioè la necessità di costruire strumenti che obblighino, laddove questa cooperazione non si produca spontaneamente, gli attori del territorio o della situazione produttiva in analisi a una cooperazione positiva, al fine di prevenire i rischi derivanti dalla complessità. Siamo in un mondo in cui la complessità del ciclo produttivo è destinata ad aumentare, anche in ragione dell'intervento di nuove tecnologie, spesso non comprese da tutti gli attori del contesto. Su questo punto è necessario sperimentare pratiche a cui probabilmente potranno seguire interventi normativi. Il nostro primo primo obiettivo non è stato quello di legiferare ancora, ma di offrire elementi concreti di riflessione, utili anche per i contesti locali. Spero di cuore - ma su questo sono ottimista - che il Governo vorrà e potrà far tesoro di questo contributo

È un'attività per conoscere, prevenire e affrontare un flagello della nostra società, quello degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, che purtroppo continua a manifestarsi in tutta la sua gravità, con incidenti quotidiani, spesso con esito mortale. Un triste fenomeno al quale non ci possiamo rassegnare, che deve trovarci tutti uniti, al di fuori degli schieramenti politici, per una battaglia che può e deve portare a ridurre al minimo, magari un giorno ad azzerare, il numero di coloro i quali escono di casa al mattino per svolgere il proprio lavoro e non fanno più ritorno dalle loro famiglie. Solo per ricordare alcuni degli eventi più gravi di questi ultimi mesi: l'incidente occorso presso la stazione di Brandizzo del 30 agosto dell'anno scorso, nel quale hanno trovato la morte cinque lavoratori; poi Firenze, il 16 febbraio scorso, dove per il crollo di una trave all'interno di un cantiere hanno perso la vita cinque operai; ancora, l'esplosione della centrale idroelettrica di Bargi, con il decesso di sette persone; l'esplosione alla Toyota di Bologna della scorsa settimana, con la morte di due giovani lavoratori; ancora, la giovane guardia giurata, Nicolò Meloni, deceduto per il crollo di una cancellata sabato scorso, ventesima vittima sul lavoro in Sardegna nel 2024. Come non ricordare la tragica fine di Satnam Singh, bracciante indiano che, invece di essere soccorso, era stato abbandonato davanti alla sua abitazione con il braccio tranciato, poggiato su una cassetta utilizzata per la raccolta degli ortaggi e poi deceduto a seguito delle gravi ferite, e i tanti, troppi infortuni che funestano quotidianamente le cronache nazionali, mettendoci di fronte alle nostre coscienze. Non può sollevarci la recente relazione dell'INAIL, che mostra come il numero delle denunce di infortunio nel 2023 abbia registrato, rispetto all'anno precedente, una diminuzione sia dei casi nel complesso, sia degli infortuni mortali. Infatti, le denunce rilevate sono state oltre 590.000 cento rispetto alle 704.000 del 2022), di cui 1.147 con esito mortale, con una diminuzione del 9,5 per cento rispetto al 2022. Un tragico bollettino di oltre tre morti al giorno sul lavoro. Come Come ha affermato il presidente Mattarella all'indomani dell'ultima tragedia di Bologna, non ci sono più parole adeguate per esprimere l'allarme e l'angoscia. Ci troviamo di fronte ad una vera emergenza, un intollerabile fenomeno non differibile, una sfida che va affrontata sia con l'introduzione di interventi normativi, sia attraverso misure pratiche ed effettive, in grado di incidere sull'operatività del sistema sicurezza. La Commissione, pertanto, in questi mesi di lavoro non si è limitata a effettuare sopralluoghi nei luoghi dove gli episodi si sono verificati, ma fin dal principio della sua attività ha operato in una prospettiva nuova, che comprendesse, oltre all'analisi delle situazioni, anche l'elaborazione di concreti strumenti di intervento per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Un approccio diverso da quello tradizionalmente utilizzato, non solo di ascolto dei soggetti coinvolti nelle diverse realtà studiate, ma anche mirato ad elaborare soluzioni in collaborazione con le prefetture, considerate il corretto punto di coordinamento e di raccordo di tutte le istituzioni coinvolte nella raccolta dei dati e delle problematiche relative alla sicurezza del lavoro. Un'attività innovativa, che si prefigge lo scopo di sviluppare strumenti di concreto intervento, per migliorare il sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro, percorrendo la strada del confronto e dell'elaborazione di un progetto condiviso con tutte le istituzioni, specie quelle preposte ai controlli. A tal proposito costruttivi sono stati gli incontri che la nostra Commissione ha avuto con l'analoga commissione della Regione Lombardia e con i componenti del Consiglio comunale di Milano, utili per raccogliere indicazioni di buone pratiche, sulla base di esperienze positive ottenute in quei territori, che possono rappresentare meccanismi di successo perché basate su uno stretto coordinamento fra le attività dei diversi soggetti istituzionali e la collaborazione con le parti sociali. Proprio in questo contesto si sta sviluppando una convenzione della Commissione con il dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, per elaborare un progetto di studio e intervento atto a migliorare la prevenzione e la sicurezza. Basandosi su questo supporto e sull'esperienza di questi casi positivi, la Commissione si è proposta di elaborare e diffondere delle linee guida, un vero e proprio decalogo della prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro, per sperimentare l'efficacia nei vari contesti lavorativi anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, soprattutto in quelle situazioni dove più vi sono state più carenze e nei luoghi più fragili. C'è la consapevolezza che per ottenere dei risultati concreti è necessario il coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate, quindi il Ministero del lavoro, quello della salute e di tutti gli organi di vigilanza, nonché delle parti sociali e del terzo settore. Infine, è della massima importanza la diffusione delle linee guida nelle scuole e nelle università. Un altro aspetto che è emerso dai lavori della Commissione è il rilancio dell'apprendistato e della formazione duale, pensati come una fase formativa fondamentale che non deve limitarsi all'acquisizione della professionalità *(Applausi)*, ma deve anche avere una specifica una specifica attenzione alla cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Vorrei evidenziare ai colleghi come la sicurezza del lavoro è stata e sarà una priorità dell'azione del Governo Meloni, a partire dal confronto costante tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese, che è indispensabile per diffondere la cultura della prevenzione in uno sforzo comune. Una strategia, quella del Governo, basata su più prevenzione, più controlli e pene più severe per chi non rispetta le regole. Ricordo a tal proposito l'assunzione di nuovi 1.600 ispettori del lavoro (quindi un aumento considerevole del numero delle ispezioni). la patente a crediti, operativa dal 1° ottobre per il settore dell'edilizia, che ha già raccolto un'adesione molto importante delle imprese; è una novità che non solo monitora, ma incentiva il miglioramento dei livelli di sicurezza nei cantieri, perché premia le imprese virtuose e sanziona quelle che non rispettano le regole. Il Governo è intervenuto anche sulle sanzioni, sia amministrative che penali, reintroducendo il reato di somministrazione illecita di lavoro, una fattispecie depenalizzata in passato, ma che risulta essere la più cresciuta nel tempo. Maggiori risorse sono state destinate per i bandi ISI, uno strumento importante per incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori delle micro e piccole imprese nel settore agricolo, con un finanziamento che è passato da 333 a 500 milioni nel 2024. Ricordo poi la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni per studenti e personale delle scuole di ogni ordine e grado. Sono tutti segnali importanti che mostrano l'attenzione che il Governo sta ponendo su questa drammatica emergenza; una sfida che, in primo luogo, non può che essere culturale, a partire dalle istituzioni scolastiche, per formare i cittadini e fare in modo che siano consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele dei lavoratori. Concludo, colleghi, riportando le parole della Presidente del Consiglio in occasione della recente relazione all'INAIL. La sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un diritto di ogni lavoratore; garantire questo diritto è una priorità permanente che deve vedere tutti in prima fila.

a firma di senatori rappresentanti dei Gruppi parlamentari, il cui testo è in distribuzione. Ha facoltà di parlare il relatore.

se saremo in grado di discutere tra noi mettendo al centro prima di tutto i diritti della persona e quindi dei lavoratori e delle lavoratrici, credo che saremo in grado di dare una risposta positiva in questa direzione. Saranno poi i fatti a darne dimostrazione. Noi vorremmo in sostanza che

Ovviamente l'obiettivo è arrivare a morti zero, però in questo caso bisogna davvero fare uno sforzo per dare un colpo di reni e abbattere fortemente questi drammi, che, dal punto di vista sia personale che economico e sociale, sono un dramma per tutto il Paese. I costi umani e i costi economici sono infatti rilevantissimi per questo sono d'accordo con chi sottolineava che investire sulla sicurezza è un fatto positivo,

Grazie,

Durigon, che oggi sostituisco; ciò in qualche modo vede entrare anche il Ministero dell'interno in quella interconnessione di cui parlava il relatore rispetto alle prefetture, che diventano un punto importante di confronto. un tema che credo non veda assolutamente divisioni e che va risolto. Chi, prima di arrivare in queste Aule, ha amministrato per tanti anni la cosa pubblica e gli enti locali, gestendo cantieri, credo che non sia stato immune, purtroppo, da qualche tragico episodio di chi

farne una questione culturale. Non è un costo, ma è un investimento, quello della sicurezza. È necessario anche utilizzare l'intelligenza artificiale in modo intelligente, come in questo caso.

Mi affido al Presidente, per il futuro, perché non ci si ritrovi in Aula a dover prendere atto di contenuti che magari possono essere comunicati preventivamente e su cui c'è la possibilità di dare un nostro consenso in maniera pragmatica.

formalmente i diritti dei lavoratori; un complesso di norme oggetto nel tempo anche di interventi legislativi, ma che segna sicuramente l'inizio o quantomeno l'esordio della consapevolezza del diritto del lavoro e dei lavoratori al rispetto delle loro condizioni sancite già nella Costituzione, che impegna e riconosce il diritto dei lavoratori ad avere un ambiente di lavoro che ne tuteli l'integrità psicofisica e la dignità come persone. I riferimenti normativi quindi sono importanti; come dice il presidente Mattarella, la Costituzione non afferma, riconosce un diritto e, nel momento in cui lo riconosce, significa questo diritto già esiste, è qualcosa che è immanente. Il compito del legislatore, allora, nel momento in cui il diritto è riconosciuto, è tutelarlo.

una lacuna che andrebbe colmata anche con un'opportuna deroga; non si può costituire una Commissione di inchiesta così importante e lasciare fuori un Gruppo dai suoi lavori, anche per le conseguenze che abbiamo visto con la presentazione di una proposta di risoluzione di cui abbiamo preso conoscenza soltanto in Aula, senza che questo costituisca assolutamente, presidente Magni, un rimprovero nei suoi confronti; sto parlando in senso generale. Ho apprezzato molto l'esposizione, ho letto anche la relazione presentata dalla Commissione, di cui chiaramente condivido il contenuto e il senso del lavoro svolto con grande accuratezza, con grande coscienza, con la volontà dichiarata ed espressa che trova una chiara manifestazione nel testo della relazione di volere davvero risolvere questo dramma - perché questo è - delle morti e degli infortuni sul lavoro, che vanno purtroppo crescendo. Il *trend* in crescita rispetto al 2023 segnala un aumento del 3,5 per cento. Questi non sono numeri o, meglio, i numeri in questo caso più che mai ci devono fare capire che dietro di essi ci sono le persone e dietro le persone ci sono i drammi, ci sono famiglie che perdono propri familiari, spesso giovani, come nel caso dello stabilimento della Toyota a Bologna, con due operai giovanissimi che hanno lasciato famiglie nello sconcerto e nel dolore più grande. Lo stesso è accaduto purtroppo negli altri incidenti mortali sul lavoro che ci sono stati nel corso dell'ultimo anno, di cui spesso abbiamo fatto nell'Aula del Senato una commemorazione sentita e partecipata da parte di tutti noi. Il dramma della morte sul lavoro è inconsolabile perché avviene nell'ambito in cui, come dice sempre la nostra Costituzione, l'uomo esprime se stesso. Il cittadino italiano ha un diritto e un dovere a lavorare e nel lavoro la Repubblica riconosce i suoi fondamentali, i suoi principi più importanti. Morire sul luogo di lavoro è come morire nel momento in cui si contribuisce alla Nazione. È una perdita non soltanto individuale, ma per tutti noi, per lo Stato, per la Nazione, per l'Italia. È una perdita di fronte alla quale noi, come legislatori, oltre a fare un'inchiesta e indagarne le ragioni, dobbiamo necessariamente interrogarci su cosa si possa fare per migliorare questa condizione e sulle ragioni per le quali gli strumenti che fino ad ora sono stati

Questa domanda non ci deve impegnare semplicemente in maniera formalistica, dicendo che noi più di quello che abbiamo fatto, non possiamo fare. Al contrario, fintanto che l'obiettivo non verrà raggiunto, significa che la responsabilità è condivisa, che qualcosa non funziona e che noi non riusciamo a capire che cosa. Su questo punto la relazione ci fornisce strumenti di riflessione sui quali però è necessario fare un ulteriore approfondimento,

e di attenzione da parte dei lavoratori più grandi, che forse anche per un retaggio culturale sottovalutano gli aspetti della formazione o, forse, non hanno sviluppato, a causa sempre di un retaggio culturale che vuole il lavoratore quasi un beneficiario di una prestazione e della sua retribuzione, lo vuole un po' sottomesso, un po' timido, poco propenso a rivendicare il rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Prova ne sono gli incidenti che si sono verificati, gravemente spesso annunciati e già molte volte oggetto di rivendicazioni da parte delle organizzazioni sindacali che denunciavano l'assenza di condizioni di sicurezza, che preannunciavano quelle che purtroppo sono state delle stragi che si dovevano evitare. Quanto più succede questo, tanto più vuol dire che il modello organizzativo di quell'azienda è un modello errato. E non ci può neanche star bene quello che è accaduto a Bologna dopo la strage, perché la vicenda di un *boiler* che esplode all'esterno, rompe la parete e uccide i lavoratori all'interno non si può concludere certamente con la messa in cassa integrazione di tutti i lavoratori. Non ce ne possiamo lavare le mani così,

per la considerevole quota del triplo rispetto ai lavoratori italiani; anche questo significa che c'è un *deficit* di formazione, ma soprattutto di consapevolezza. Un ultimo accenno lo voglio dedicare alla patente a punti; sempre le statistiche ci dicono che i tre ambiti nei quali gli incidenti mortali sono più diffusi sono l'edilizia, l'agricoltura e il settore manifatturiero e nell'edilizia il Governo ha pensato di introdurre la patente a punti, che poi sostanzialmente è una sorta di certificazione-a credito: si parte con il massimo del punteggio e se si mantengono gli *standard* o si fanno investimenti sulla sicurezza e se non si verificano infortuni o incidenti, il punteggio va aumentando. Questo, però, è uno strumento di partenza che, come tutte le autocertificazioni, come tutto ciò che viene dato preventivamente per buono, implica che poi si debbano fare investimenti sui controlli e soprattutto si debbano adottare misure severe

una riflessione ancora più approfondita, perché quando gli ispettori del lavoro si recano in un cantiere e trovano dei lavoratori che lavorano in nero, scattano immediatamente le sanzioni che prevedono una sanzione pecuniaria molto importante e l'obbligo di assunzione. Benissimo, ho sentito dire che, a seguito dei controlli, sono state fatte soprattutto nell'ambito dell'agricoltura notevoli assunzioni, ma questo di per sé è un dato che ci dice ben poco, perché la realtà e l'esperienza ci dicono che queste aziende, dopo avere assunto, probabilmente poi licenzieranno tutti, perché non riusciranno a mantenere questo carico, questa spesa. Questo significa che si combattono gli infortuni sul lavoro e si fa veramente un investimento imponendo, quando si fanno appalti, quando si danno lavori, quando si fanno le verifiche, che il carico assunzionale di un'impresa sia parametrato all'entità del lavoro che deve svolgere, perché se noi continuiamo ad aggiudicare lavori a ditte che hanno cinque operai per fare il lavoro che dovrebbero fare in 25, è chiaro che poi il costo di questa riduzione del personale si

che la presiede per le cose che ci ha detto stamattina, per il suo, secondo me, molto giusto intervento e naturalmente anche per il lavoro che la Commissione ha svolto in tutti questi mesi, per le tante missioni che ha svolto e per questa risoluzione, per l'appunto, che mi sembra

della sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui stiamo parlando, in maniera concreta e pragmatica, per esempio cercando di far diventare la prevenzione l'anello attorno al quale far ruotare il lavoro politico e naturalmente anche un intervento legislativo che poi si dovrà fare e anche immaginando delle vere e proprie sperimentazioni, chiamiamole così, di un nuovo metodo di lavoro che pure io penso possa essere particolarmente utile. Insomma, mi sembra un contributo reale per provare ad intervenire concretamente Il senatore Magni l'ha detto molto bene e ha spiegato con parole molto chiare, illustrando oggi il lavoro fatto in questi mesi dalla Commissione e centrando la sua attenzione su un punto che anche a me pare particolarmente rilevante. Mi riferisco a quello che egli ha definito la mancanza,

materia, intervenire non dentro una dimensione collettiva, ma - invece - singolarmente e, quindi, senza quella necessaria sinergia che noi riteniamo invece decisiva e fondamentale. Il protocollo che viene

dei risultati. I dati li conosciamo, sono stati spiegati bene nel corso della discussione di stamattina. Ne hanno parlato adesso la senatrice Musolino e qualche minuto fa la senatrice Tajani. È evidente che siamo dinanzi a una condizione che non ha visto un miglioramento nel corso di questi anni, ma anzi - purtroppo - un peggioramento. I dati ci dicono che in Italia continuano a morire più di tre lavoratori al giorno. La morte recentissima dei due operai alla Toyota di Bologna, venerdì 25 ottobre, è solo l'ultimo caso cui è stato dato risalto dalle cronache nazionali. Anche le denunce di infortunio sono molto aumentate: 351.000 sono quelle riguardanti i primi sette mesi del 2024, in aumento dell'1,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche le denunce di infortunio con esito mortale presentate nei primi sette mesi del 2024 sono più di quelle registrate nello stesso periodo del 2023.

più ampia e trasversale possibile, un'analisi più approfondita del contesto e forse anche una maggiore necessità di confronto a livello nazionale sul tema della sicurezza.

altrettanti fenomeni di grande rilevanza e anche preoccupazione che non sono mappati come dovrebbero. Si pensi, tanto per dirne uno, allo sfruttamento

in questi ultimi anni di crisi economica. In Italia si stima che siano oltre 300.000 i minorenni, che dai sette ai quindici anni hanno avuto esperienze

Una parte significativa - uno su tre - ha svolto lavori particolarmente dannosi per i percorsi educativi e per il benessere psicofisico e naturalmente questo la dice lunga. Altra grande questione è il lavoro irregolare. Sono tre milioni le persone che lavorano irregolarmente. Insomma, si potrebbe fare un lunghissimo elenco, come sappiamo e come tante volte abbiamo detto. Ecco, io spero che la giornata di oggi possa essere l'inizio di un percorso politico importante, nuovo quindi davvero sono molto felice di poter salutare il fatto che questa risoluzione sia stata firmata dai Capigruppo di tutti i Gruppi parlamentari e di poter annunciare

almeno questo è l'auspicio, e all'unanimità si continuerà a seguire il lavoro di questa Commissione. Mi permetta innanzitutto di evidenziare l'ottimo lavoro che la Commissione d'inchiesta ha svolto sotto la presidenza del senatore Magni. Anche per noi l'impegno sul territorio, nei luoghi di lavoro, nella comprensione dei fatti e degli accadimenti, perché si potesse intervenire con le risposte più adeguate, credo che sia la direzione giusta e l'auspicio è che si continui a lavorare in questo modo, perché la Commissione sta davvero svolgendo un importante impegno. importante impegno. Sul territorio sta entrando nei meccanismi delle migliori pratiche da adottare e negli ambienti di lavoro sappiamo quante variabili ci siano e quante variabili portino poi a diverse interpretazioni, a dover capire quello che accade, come accade e come si può evitare - perché questo è l'auspicio - il ripetersi di incidenti in cui troppo spesso nostri concittadini perdono la vita. È già stato detto che perdere la vita sul luogo di lavoro è davvero una cosa inaccettabile. Ci uniamo anche noi all'appello affinché davvero tutto ciò che potrà essere fatto, non solo evidentemente dalla politica, dal legislatore, ma da tutte le parti sociali e da tutti coloro che rientrano nei meccanismi che rendono possibile aumentare la sicurezza sul lavoro, Condividiamo l'idea di arrivare oggi a questo atto di indirizzo comune intermedio, chiaramente continuando a fare in modo che gli atti di questa Commissione trovino un'unanimità di lavoro, di impegno e quindi anche nelle conclusioni.

che inducano le imprese all'adozione delle migliori pratiche. Il Gruppo Forza Italia continuerà a collaborare con il massimo impegno all'interno della Commissione e all'interno di tutti gli organismi che potranno contribuire al miglior lavoro di questa Commissione. Nel frattempo, oggi, come abbiamo già detto, diamo il nostro

che ci dà l'indirizzo giusto da percorrere: una collaborazione, una non strumentalizzazione di ciò che ci accade attorno per fare in modo che tutto ciò che vediamo, tutto ciò che purtroppo deploriamo,

Signor Presidente, oggi è al voto la risoluzione sull'attività svolta finora dalla Commissione d'inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia, impegnata sul dramma dello sfruttamento e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

stesso periodo dell'anno scorso. Questo significa che ci troviamo davanti a un fenomeno che presenta e merita una profonda riflessione e azioni più che mirate, concrete e e condivise. Troppe disgrazie continuano a consumarsi in un luogo che dovrebbe aiutare gli individui a vivere meglio, a donare dignità e sostentamento; invece da troppo tempo è sinonimo anche di pericolo.

Non è quanto ci si dovrebbe aspettare in un Paese industrializzato nel 2024, con tutele strutturate e sistemi di prevenzione accreditati. Nei fatti tutto dovrebbe essere perfetto, ma invece resta mera teoria. I settori investiti da queste denunce mortali sono molteplici, troppi: si va dal comparto edilizio a quello manifatturiero, dall'agricoltura ai trasporti. Gli infortuni sul lavoro non solo impattano gravemente sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie, ma costituiscono anche un danno economico rilevante per lo Stato. Basti pensare che, secondo stime recenti dell'INAIL, il costo complessivo degli infortuni e delle malattie professionali ha superato i 50 miliardi di euro annui, pari a circa il 3 per cento del PIL nazionale. Questi dati impongono un intervento perentorio e non più procrastinabile. La sola repressione non è sufficiente, come abbiamo detto tutti; occorre puntare su prevenzione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori. Questi temi sono costantemente presenti nei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta di cui faccio parte. Colgo l'occasione per rivolgere un plauso al presidente Magni, che ha condotto, sempre con la massima condivisione e attenzione, i lavori della Commissione. Ringrazio anche tutti i colleghi per essere sempre attivi su una tematica e un impegno comuni. Lo studio dei fenomeni e la loro analisi è di strategica importanza: con questa consapevolezza abbiamo condotto anche diverse missioni da Nord a Sud, con l'ambizione di proporre strumenti di intervento concreti, e quindi dare una sferzata di innovazione al composito sistema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Investire in questo campo non è solo un imperativo che mette in gioco etica e morale, ma anche un piano concreto che genera effetti positivi. Quando le aziende scelgono di investire in prevenzione, i sinistri e le gravità delle lesioni si abbassano. Quando si dà più dignità ai lavoratori, trattandoli come parte essenziale e preziosa del progetto produttivo, anche la redditività migliora, migliorando l'aspetto psicologico del singolo e dell'intero ambiente lavorativo. Tuttavia, tutto questo non può rappresentare una questione in cui è coinvolta una sola parte; la responsabilità non può essere unilaterale. È necessario coinvolgere tutti i soggetti interessati, aziende e associazioni di categoria, enti locali e naturalmente, *in primis*, lo Stato in tutte le sue diramazioni, per le giuste giuste interconnessioni. «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»: così recita l'articolo 4 della nostra Costituzione. Questo diritto però non può e non deve trasformarsi in una sentenza di morte. Lo Stato infatti deve creare le condizioni affinché tutti abbiano le stesse opportunità per trovare occupazione e, nello stesso tempo, impedire che questo prezioso strumento di emancipazione sociale assuma le sembianze di una pistola puntata alla tempia, pronta a sparare al minimo contrattempo. A questo proposito, è altrettanto importante fare informazione sugli eventi cosiddetti quasi incidenti. Si tratta di campanelli di allarme, di piccoli segnali oppure, più spesso, di grandi segnali, che non devono assolutamente essere trascurati. Parliamo di episodi che non hanno comportato effetti gravi per una serie di concomitanze propizie, ma che hanno tutto il potenziale per diventarlo. Tenere traccia di questi fenomeni e analizzarli vuol dire scongiurare potenziali pericoli e difendere concretamente la salute dei lavoratori. Anche l'indicazione dei casi di successo sperimentati ha la sua valenza, perché significa coinvolgere sinergicamente le situazioni virtuose. È quello che abbiamo fatto proprio nelle fasi iniziali dell'attività di inchiesta portata avanti dalla Commissione. La conoscenza dei concetti portanti della sicurezza sul lavoro è un altro punto centrale. La sicurezza non deve essere raccontata e interpretata dall'esterno come una noiosa osservanza normativa, ma deve essere percepita come un valore necessario e basilare nell'organizzazione aziendale. Per promuovere questo cambio di mentalità è necessario diffondere questa cultura già dai primi anni di scuola. In tal senso, credo fermamente nell'integrazione di programmi di educazione alla sicurezza nel sistema scolastico, perché ogni giovane possa essere sensibilizzato al rispetto delle norme di sicurezza come futuro lavoratore e auspicabilmente futuro datore di lavoro. Dunque formazione continua per una radicata cultura della prevenzione e adozione delle buone pratiche in ogni ambito lavorativo. La nostra responsabilità come legislatori è di costruire un sistema di regole che non solo protegga i lavoratori, ma che incoraggi operosamente un ambiente di lavoro più sicuro, rispettoso dei diritti e sostenibile per le generazioni future. È un impegno che dobbiamo assumere senza riserve, poiché la sicurezza non è un costo, ma un investimento essenziale per il benessere di tutti. che oggi ci apprestiamo a votare è frutto di un lavoro condiviso e unanime, senza colori politici - l'abbiamo detto - e senza nessun costrutto preconfezionato o barriere ideologiche. Il sentire prevalente, infatti, è quello della difesa assoluta e totalizzante dei lavoratori. Sviluppare un indirizzo unitario vuol dire dare concretezza all'azione che si svolge in Commissione, partendo dall'ascolto di chi opera negli svariati ambiti e facendo tesoro delle soluzioni proposte e delle iniziative virtuose assunte. Un lavoro teso all'elaborazione di strumenti di intervento volti a migliorare il sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro, percorrendo la via della concertazione e dell'elaborazione condivisa con le istituzioni preposte ai controlli. In particolare, la Commissione ha fatto leva sulle funzioni di coordinamento delle prefetture, che costituiscono un prezioso punto di riferimento sia per i dati raccolti, sia per la conoscenza dei fattori critici, oltre a essere la sede più opportuna per l'elaborazione di protocolli efficaci. Il coordinamento e la collaborazione trovano terreno fertile laddove vi sia condivisione di dati, di proposte e di risultati e dove vi sia l'apertura su questioni nuove e possibili soluzioni. Pensiamo all'intelligenza artificiale: anche lì la nostra attenzione è molto precisa a individuare i vari aspetti di utilità per la soluzione di queste problematiche. Resta ferma e concreta, oggi, la necessità di migliorare le condizioni di lavoro; è evidente dai dati funesti e dalle denunce. È necessario disincentivare comportamenti di intermediazione illecita e di sfruttamento. Anche questo è un punto rilevante, che è stato più volte sollecitato e sottolineato dai colleghi, perché più aumentano gli appalti e i subappalti e più aumenta il rischio di questi eventi. A questo riguardo, risulta incisivo lo strumento della piattaforma di filiera, attraverso la quale viene messa in chiaro la profilazione delle imprese e della manodopera impiegata. C'è da dire che c'è ancora tanto da fare. Siamo sulla strada giusta e non dobbiamo demordere, ma, al contrario, essere più convinti che mai che la cultura della sicurezza sul lavoro è una conquista a cui deve mirare l'impegno di tutti. Per questa ragione annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. io non entrerò molto nel merito di quello che è il lavoro fatto dalla Commissione e, quindi, della relazione intermedia. Mi limito solamente ai ringraziamenti in questo senso al Presidente e a tutti i componenti della Commissione, agli Uffici, alla parte amministrativa e alla parte tecnica. Ritengo importante sottolineare come questa Commissione abbia intrapreso un lavoro innovativo, ma soprattutto pragmatico e concreto. Complimenti davvero per la relazione. Vorrei soffermarmi invece sul provvedimento che siamo chiamati a discutere e votare. Una soluzione che ci tocca, come hanno detto tutti i colleghi, nel profondo poiché riguarda un tema di grande importanza, la sicurezza nei luoghi di lavoro di lavoro e - tengo a sottolineare questo che è un aspetto importante - i percorsi di formazione e lavoro. In questo mio intervento non posso non ricordare Lorenzo Parelli, un giovane studente dell'Istituto Bearzi di Udine, dalla Regione da cui provengo che purtroppo ha perso la vita proprio nell'ultimo giorno di lavoro del suo percorso di scuola lavoro, in un tragico incidente avvenuto in una fabbrica, per il quale le condanne che sono state fatte in questi giorni non gli restituiranno la vita. La sua storia drammatica e ingiusta non è e non deve essere solo un monito per noi, ma anche un richiamo a quella che viene definita nel documento che noi abbiamo presentato, una responsabilità collettiva. Da quel tragico episodio è nata, lo sapete, la Carta di Lorenzo, un documento che stabilisce quelli che sono i principi essenziali per la sicurezza e la tutela dei giovani che sono impegnati nei percorsi di formazione lavoro. Questa Carta si propone di fissare regole molto chiare, vincolanti, che pongano al centro il diritto alla sicurezza e la responsabilità di tutti quelli che sono gli attori coinvolti. In questo senso mi riferisco agli enti formativi, alle aziende e, naturalmente, alle istituzioni, quindi anche a noi. Troppe volte negli ultimi anni abbiamo assistito ad incidenti sul lavoro che hanno coinvolto anche giovani in formazione, ragazzi che entrano nelle nostre aziende con entusiasmo e speranza per il proprio futuro e, poi, evidentemente ne escono con una drammatica soluzione come quello che è accaduto a Lorenzo. Oggi, attraverso il voto di questa importante risoluzione, abbiamo davvero l'occasione di onorare non solo la sua memoria, ma anche quella delle tante vittime sul lavoro che attraverso azioni concrete, rafforzando quelle che sono le misure di sicurezza, sviluppando strategie innovative e più stringenti percorsi formativi, consentiranno di diminuire quel drammatico incremento delle morti sul lavoro a cui costantemente siamo costretti ad assistere. È quindi una nostra responsabilità garantire che chi si avvicina, soprattutto i giovani, al mondo del lavoro non venga esposto a rischi che evidentemente sono evitabili. Gli studenti, in particolare, devono essere accompagnati, formati e seguiti da professionisti consapevoli della delicatezza del loro ruolo in un ambiente che rispetti le normative sulla sicurezza e valorizzi la vita umana al di sopra ogni altra esigenza. Probabilmente se mi fossi trovato nell'altro emiciclo dell'Aula, avrei detto profitto. La Carta di Lorenzo, rappresenta allora un passo in avanti in questa direzione, ponendo l'accento sulla necessità di un'alleanza educativa tra scuola e lavoro che non scarichi sui giovani la mancanza di mezzi e di risorse, ma formi cittadini che saranno poi i lavoratori di domani, consapevoli soprattutto di quelli che sono i rischi che ogni professione comporta. Il lavoro quindi deve essere un'opportunità di crescita e non un campo di battaglia, specialmente per i nostri giovani; ogni incidente mortale è un fallimento delle istituzioni, un grido di dolore che noi non possiamo e non vogliamo ignorare. Per questo nella risoluzione che oggi voteremo sosteniamo l'introduzione - e questo e questo è un passaggio fondamentale - di un progetto e una sperimentazione attraverso protocolli efficaci, linee guida contestualizzate, analisi e sviluppo di buone prassi, ma anche percorsi di formazione continua per tutti i soggetti coinvolti, dalle aziende ai lavoratori, agli insegnanti, ai *tutor* finanche agli studenti. La sicurezza deve diventare un elemento fondante della cultura scolastica lavorativa, un principio su cui noi non possiamo assolutamente accettare compromessi. Voglio concludere omettendo una parte della mia relazione, perché molte delle cose che mi sono appuntato sono state dette dai colleghi e quindi la lascerò agli atti, atti, ma sottolineando che oggi abbiamo una grande opportunità, che è quella di prendere una posizione chiara e decisa e non possiamo assolutamente permetterci di fallire. Ogni nostra decisione, ogni voto che andremo ad esprimere incide sulla vita di chi ci osserva e sono tutte persone che si affidano con grande fiducia al nostro lavoro, al lavoro delle istituzioni. Facciamo allora in modo che il nostro impegno sia davvero un segnale forte per tutte le famiglie, per tutti i lavoratori e per tutti i giovani, ma io direi per tutta la nostra comunità. La sicurezza sul lavoro è un diritto e una responsabilità che noi non possiamo delegare a nessun altro e soprattutto non possiamo trascurare.

di far parte di una Commissione che ha visto in questo ramo del Parlamento, per molti anni, la direzione da parte di Luciano Lama. è tra coloro che hanno portato il tema della sicurezza sul lavoro dall'essere una questione interna ai luoghi di lavoro, limitata al rapporto tra i lavoratori e le aziende, a essere anche un grande fatto normativo, una questione che richiama la responsabilità di tutti. Cosa che è avvenuta - e Luciano Lama ben rappresentava tutto questo - quando è cambiata la cultura stessa; chi tra di noi ha qualche anno di più si ricorderà quando la salute nei luoghi di lavoro veniva o monetizzata, dando per scontato che non era possibile prevenire i danni derivanti dalle condizioni di lavoro, quindi si preferiva pagarla, oppure risolta dal fatto che si prendevano delle sostanze e si sperava che evitassero le conseguenze. Quando si prende coscienza di sé, della relazione tra il proprio corpo e il proprio essere e le sostanze e i luoghi di lavoro, le temperature, le posizioni, è lì che sulla sicurezza sul lavoro si fa uno straordinario salto di qualità, perché si scopre che è davvero possibile prevenire. Non c'è solo il problema di risarcire rispetto alle conseguenze, ma il valore della vita dei lavoratori e delle lavoratrici e della loro buona salute, della loro buona condizione viene messo a premessa. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro nel proporre un ragionamento connesso a buone pratiche e a *governance*, esattamente perché assumiamo quel principio. Il compito della Commissione, come della politica non può essere quello di accorgersi della questione sicurezza sul lavoro ogni volta che piangiamo un lutto, perché se ci siamo solo quando c'è da commemorare vengono in mente più le lacrime di coccodrillo che non la responsabilità della politica ad affrontare i problemi. *(Applausi)*. Non si può essere essere responsabili solo nella ricerca delle parole giuste nelle purtroppo frequenti occasioni in cui dobbiamo piangere uno o più morti negli incidenti che si susseguono. La responsabilità è provare a tradurre nella quotidianità, nell'oggi e nel cambiamento cosa vuol dire assumere quel tema del benessere della condizione dei lavoratori e delle lavoratrici che pure nella storia che abbiamo alle spalle ha fatto tanti salti di qualità. Il tema non è solo Il tema non è solo dirci responsabili, ma è come traduciamo quella responsabilità, perché dirci responsabili è essenziale e semplice. la Sottosegretaria presente, ma non posso non rammaricarmi dell'assenza del Ministro del lavoro in questa occasione. Non sono tante le occasioni in cui le Camere si riuniscono per discutere di che cosa fare specificamente su questo tema e per presentare anche un rapporto di lavoro e forse sarebbe stata un'occasione utile per esserci, anche perché credo che la discussione su questo insegna a tutti voi e a tutti noi degli elementi che sono importanti. Vorrei andare a fondo del tema che è stato citato da tutti i colleghi e le colleghe intervenuti. Dobbiamo produrre cultura della sicurezza sul lavoro ed esercitare quella responsabilità, da un lato - lo abbiamo detto, come Commissione - attraverso processi di *governance* e impegno dei soggetti e, dall'altro, diffondendo e disseminando cultura della sicurezza sul lavoro. Credo sarebbe bene se provassimo a esercitarci davvero, così come facciamo in Commissione, sul tema della cultura della sicurezza sul lavoro. Cultura della sicurezza sul lavoro non è solo piangere e inchinarci di fronte ai grandi incidenti, ma è anche domandarsi che cosa sta succedendo concretamente nei luoghi di lavoro quando alcune cose sono profondamente cambiate. Possiamo dire che spesso la reazione rispetto al tema della sicurezza del lavoro è a posteriori, quando si verifica l'incidente, il che vuol dire che i lavoratori sono meno forti nella capacità di denunciare e prevenire quelle condizioni. Interroghiamoci sul perché sono meno forti, perché non c'è una capacità di prevenzione data dall'istintiva necessità che i lavoratori e le lavoratrici sappiano in quale contesto lavorano. lavorano. Anzitutto dobbiamo dire che crescono appalti e subappalti e, quindi, aumentano i luoghi in cui è difficile, anche perché magari non si conosce dove si sta andando a lavorare, non si conoscono coloro che lavorano intorno a sé e insieme a sé, non si conosce qual è complessivamente l'opera che si sta affrontando. Le colleghe precedentemente hanno citato i protocolli di anticipo - così li chiamavamo - che prevengono le possibili difficoltà durante le grandi opere. Tuttavia, è difficile che anche quel protocollo regga fino in fondo se poi i lavoratori tra loro non si conoscono e se ci sono lavoratori che si trovano in condizione di solitudine e nell'impossibilità di avvisare se hanno dei problemi. Dobbiamo dircelo: i lavoratori fanno più fatica a proteggersi rispetto a condizioni di non sicurezza, perché la precarietà è un indebolimento della loro possibilità di reagire e rifiutarsi se ci sono condizioni. Cultura della sicurezza è anche sapere qual è il rapporto di lavoro e che possibilità hanno i lavoratori. È un punto di sicurezza e di possibilità o meno di esercitare la propria capacità di scegliere. Bisognerebbe anche cominciare a parlare delle malattie professionali, perché anch'esse sono connesse ai processi di prevenzione. Sapere che sostanze si usano, se quelle sostanze vanno sostituite ed evitare logiche di risparmio, invece il problema del benessere delle persone, è straordinariamente necessario. Bisogna sapere che le malattie cambiano. Lo sappiamo quando discutiamo di sanità e bisognerebbe saperlo anche quando si parla di sicurezza sul lavoro, perché cambiano i contesti, le possibilità di avere delle relazioni, perché cambia il modo di lavorare. Noi tutti siamo immersi in una grande transizione che è quella del digitale, ma in realtà non abbiamo alcuna idea di che cosa quel cambiamento determina sulle menti delle persone e, anzitutto, dei lavoratori e delle lavoratrici. Eppure, se guardiamo con un po' di attenzione a cosa sta succedendo nei luoghi di lavoro, ci accorgiamo che, per esempio, aumenta l'uso degli psicofarmaci e di forme di resistenza, di possibilità di sostanza necessaria a resistere nei luoghi di lavoro. Siamo sicuri che sia una buona pratica? Siamo sicuri che questo non denunci un problema che nella relazione con il cambiamento tecnologico c'è anche bisogno di domandarsi come ricostruiamo quel benessere dei lavoratori che è stato l'obiettivo? Come facciamo tutte queste cose, non solo in termini di singola rivendicazione, nel singolo ruolo, nel singolo luogo di lavoro e nella singola situazione specifica, ma come questo diventa un elemento di cultura? Se noi diciamo che prima ci sono la vita e la certezza delle persone, dobbiamo anche dire che ogni volta che esaminiamo un contesto, dobbiamo leggerlo anche alla luce della certezza che ci sia sicurezza sul lavoro. Dobbiamo chiedere che la progettazione dei luoghi di lavoro, dei cantieri e di tutte le situazioni venga fatta tenendo conto che c'è un tema di prevenzione e di messa in sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Provo a tradurla così: deve sparire l'affermazione, che troppo spesso si fa, secondo cui la sicurezza sul lavoro è un costo. Infatti, ogni volta che lo si affronta come costo, in realtà c'è dietro il pensiero che allora è meglio ridurlo il più possibile, perché non è vissuto come un investimento. le parole che ha detto recentemente l'amministratore delegato di una grande azienda, che forse provocatoriamente era stato interpellato. Gli era stato chiesto: ma lei non pensa che molti degli infortuni sul lavoro sono colpa della distrazione del lavoratore, Questo amministratore delegato ha risposto dicendo: la sicurezza è una responsabilità dell'azienda e una buona progettazione prevede anche di provare a prevenire possibili disattenzioni ed errori, perché noi siamo umani. E sono umani anche i lavoratori e le lavoratrici che quindi, se sono in contesti di tensione e di difficoltà - pensiamo a tutti gli elementi dello *stress* da lavoro correlato - è assolutamente evidente che può succedere, ma è nostra responsabilità che quel "può succedere" venga prevenuto. Allora lo sforzo che la Commissione sta facendo, lo sta facendo unitariamente - questa è solamente un'annotazione importante che va sottolineata - ed è questa la ragione per cui il nostro partito voterà favorevolmente alla risoluzione.

Tutti abbiamo la medesima responsabilità, quella cioè di non abusare del dolore e soprattutto di attendere ognuno al proprio dovere per fare in modo che eventi come questi non si ripetano più. Credo che la prima azione sia quella della responsabilità, che però vorrei riportare alla corresponsabilità. Nessuno può chiamarsi fuori ed ognuno può e soprattutto deve dare il proprio contributo, chiaramente in relazione al proprio ruolo. È superfluo ricordare che i problemi odierni sono il frutto di una pesantissima eredità che ormai ci trasciniamo da decenni. È fondamentale invece sottolineare che abbiamo bisogno di ricorrere a tutte le competenze per trovare soluzioni che siano oggi al passo con i tempi e che siano realmente in grado di invertire la tendenza negativa, per giungere quantomeno, se non ad azzerare, a diminuire in modo significativo il numero degli infortuni sul lavoro. In questa legislatura, dal 2022 ad oggi, l'attenzione sui temi del lavoro è sempre stata alta e si è espressa in molti provvedimenti specifici, gli incentivi all'inserimento nel mercato del lavoro e la tutela di giovani e donne - le categorie da sempre più penalizzate in termini occupazionali - la semplificazione e la razionalizzazione,

e non da ultimo con l'introduzione della patente a punti, o crediti che dir si voglia, che è sempre stata sbandierata ma che finalmente è stata messa a terra. Da un lato, i provvedimenti attuali hanno dato frutti positivi, concorrendo a determinare e consolidare un'inversione di tendenza sul mercato del lavoro in termini di stabilità occupazionale. I dati Istat lo confermano: sono dati estremamente positivi, che sono da consolidare ulteriormente, soprattutto per andare a ridurre il *gap* di cui parlavamo prima relativo alle figure, soprattutto femminili e giovanili. Dall'altro lato, invece, continua lo stillicidio degli infortuni, anche mortali, mortali, e lo si registra su tutto il territorio nazionale. Sono tragedie inaccettabili per le vittime, per i familiari, ma anche per noi che abbiamo responsabilità di governo del Paese. È qui che diventa più che mai urgente che il nostro intervento vada a incidere sulla cultura del lavoro, affinché essa si traduca in capacità di esprimere prevenzione e maggiori controlli, attraverso piani formativi adeguati, adeguati, anche all'innovazione che oggi tocca ogni comparto dell'economia, a partire dalla formazione scolastica, perché da lì tutto nasce. Occorre un sistema di controlli moderno, puntuale e flessibile, che sia in grado di disincentivare qualsiasi pratica e procedura pericolosa, e l'applicazione tempestiva delle sanzioni, atteso che la certezza della pena è sicuramente la miglior forma di deterrenza. L'attività di indagine della nostra Commissione ha preso avvio dalla conferma di una situazione emergenziale drammatica. Prima sono stati citati molti degli infortuni anche mortali che abbiamo dovuto ricordare anche in quest'Aula; sono su tutto il territorio nazionale, in ogni livello e in tutte le diverse filiere produttive; una particolare attenzione - come è già stato già detto - va all'appalto e al subappalto. L'approccio che è stato dato è alla concretezza delle risposte. Le risposte devono essere non solo adeguate alle situazioni più disparate, ma devono essere soprattutto in grado oggi di determinare cambiamenti in positivo, sia in termini di prevenzione che di moderna cultura della sicurezza. Due sono le direttrici su cui muoversi: migliorare la *governance* dei sistemi complessi, con il coinvolgimento delle diverse istituzioni - si è già detto, in particolare, delle prefetture e degli imprenditori; e promuovere ancora una volta la cultura della sicurezza, con il fine di portare al medesimo livello di consapevolezza - ribadisco, al medesimo livello di consapevolezza e di comportamenti responsabili tutti gli imprenditori quanto i lavoratori ed ogni altro soggetto che ruota intorno ai luoghi di lavoro. Quando il tema in discussione è la sicurezza delle persone occupate e l'obiettivo finale è quello della responsabilizzazione, deve innanzitutto cessare ogni forma di antagonismo. Questa è la scommessa da vincere. Questa è la resistenza da superare. Nessuno può rimanere spettatore, spettatore, perché nessuno deve lasciare ad altri decidere del proprio destino. A tale proposito, un contributo può certamente venire in soccorso dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale: a monte, nei processi iniziali di valutazione dei rischi è importantissimo nella definizione delle procedure di manutenzione; a seguire, favorendo l'automazione delle attività di *routine* e potenzialmente più rischiose; infine, attraverso il controllo mirato sulla corretta applicazione dell'esecuzione dei piani di sicurezza. A richiedere da subito un determinato livello di condivisione e corresponsione è il fattore tempo: noi non abbiamo più tempo. Il lavoro e la sperimentazione messi in atto con il Politecnico di Milano ci confermano che la strada avviata può portare ai risultati attesi. Le linee guida, ovvero il decalogo per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro, generate dall'approccio basato sulla concretezza e sullo studio delle buone pratiche in situazioni reali, saranno lo strumento guida. a condizione - come dicevo prima - che ogni soggetto coinvolto faccia la propria parte con responsabilità e consapevolezza, correlata all'importanza che assumono tutti coloro che operano nei luoghi di lavoro. Dobbiamo quindi operare con un approccio funzionale e pragmatico, rigidamente concentrato sulla definizione dei problemi e sulla loro rapida soluzione, al contrario di quello che è stato molto spesso utilizzato, ossia un approccio ideologico e disfunzionale, che definisco tale perché alla prova dei fatti non ha generato miglioramenti apprezzabili e verificabili, altrimenti non saremmo qui sempre a parlare di emergenza. Lo dobbiamo al mondo del lavoro, alle imprese e ai lavoratori, da cui ci aspettiamo molto per riportare la nostra Nazione sulla via di uno sviluppo duraturo e sostenibile. Lo dobbiamo all'Italia, alle italiane e agli italiani, che giustamente si attendono e reclamano un reale cambiamento positivo, affinché il lavoro si uno strumento di realizzazione per vivere meglio e, soprattutto, per fare in modo che di lavoro nessuno debba più morire. Sono certa che tutti faremo la nostra parte e Fratelli d'Italia farà la sua parte. Per questo annunciamo il voto favorevole su questa risoluzione.

permettetemi di esprimere il mio personale ringraziamento al presidente Magni, al vice presidente Dreosto e a tutti i senatori membri della Commissione. *(Applausi)*. Desidero ringraziarli per il grande lavoro che stanno facendo su un tema che è una vera e propria piaga sociale. Mentre eravamo impegnati in questa discussione in Aula, nel bergamasco un altro operaio di è morto, travolto da un muro in uno scavo. In sua memoria e in memoria di tutte le vittime sul lavoro e come segno di cordoglio e vicinanza a tutte le famiglie che hanno perso qualcuno mentre era al lavoro, vi chiedo di osservare un minuto di silenzio.

il caso segnalato dalla senatrice interrogante ci invita a svolgere una riflessione seria sui principi che debbono caratterizzare il processo di adozione dei libri di testo. Esso infatti rappresenta una delle fondamentali espressioni della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente garantite. Per quanto infatti, come ha riferito l'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna, il libro oggetto della presente interrogazione non risulti formalmente adottato nelle scuole primarie di quella Regione, restano valide le riflessioni svolte in questo atto ispettivo. L'adozione dei libri di testo rientra tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentito il parere dei consigli di interclasse per la scuola primaria o di classe per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, il coinvolgimento dell'intero corpo docente di ciascuna istituzione scolastica, in tal modo garantendo una puntuale verifica e un attento esame dei testi in uso, oltre che delle nuove proposte editoriali. La prima fase di valutazione dei testi rappresenta, quindi, un'occasione per la visione delle proposte editoriali da parte dei genitori rappresentanti di classe e, nella scuola secondaria di secondo grado, anche degli studenti eletti. Il criterio di fondo che presiede all'adozione dei libri di testo è definito dall'articolo 4 del DPR n. 275 del 1999, secondo il quale la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, devono essere coerenti con il piano dell'offerta formativa e attuati con criteri di trasparenza e tempestività. Inoltre, ricordo che ogni anno il Ministero per l'adozione dei testi scolastici fornisce, con apposite circolari, il quadro generale di riferimento e propone spunti ed elementi di riflessione sui vari aspetti riguardanti la materia, affinché i docenti possano effettuare valutazioni sempre più consapevoli e mirate al fine del conseguimento degli obiettivi educativi contenuti nel piano triennale dell'offerta formativa. È anche opportuno aggiungere che il libro di testo è solo uno degli strumenti, insieme a molti altri, a disposizione del docente, che se ne serve in modo libero per la realizzazione delle finalità educative e didattiche della sua azione. Ritengo comunque utile osservare che la validità didattica di un libro di testo deve essere aggiudicata all'interno delle particolari condizioni delle classi e nel contesto del piano triennale dell'offerta formativa. A tale riguardo, intendo rassicurare sul fatto che, anche per venire incontro alle esigenze rappresentate dalla senatrice, nella prossima nota per l'adozione dei libri di testo verrà ulteriormente rammentato alle istituzioni scolastiche il ruolo attivo che dovrà essere svolto dai consigli di classe e interclasse nella loro composizione allargata ai genitori e, ove previsto, agli studenti, affinché si possano effettuare valutazioni sempre più consapevoli e mirate al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi contenuti nel piano triennale dell'offerta formativa, a conferma della necessità, cui peraltro il Ministero crede fermamente del coinvolgimento attivo e consapevole delle famiglie in tutti gli aspetti del percorso formativo dei loro figli.

polemica verso il libro *gender*, ma bensì volta a porre l'attenzione del Ministero per sensibilizzare sempre di più e fare una riflessione insieme sul ruolo dei genitori come parte attiva nella scuola. Nella sua risposta, infatti, il Ministro e lei avete sottolineato l'importanza del coinvolgimento attivo e consapevole delle famiglie in tutti gli aspetti del percorso formativo dei loro figli. Bisogna andare a sensibilizzare sempre di più i genitori sulla partecipazione attiva e responsabile nelle scelte educative. La nostra società, purtroppo, sta abbandonando i nostri ragazzi a se stessi, sono loro stessi che ci chiedono aiuto e lo vediamo in diverse forme che sfociano addirittura con i famosi disturbi mentali. Non dobbiamo però lasciarli soli nel loro percorso educativo; fin da piccoli essere sempre supportati sia dagli insegnanti che dai genitori nel loro percorso di crescita verso un'educazione relazionale, nel rispetto delle persone e delle cose sia pubbliche che private. Ritengo quindi importante intervenire direttamente sull'adozione di questi libri di testo da parte dei genitori, senza intervenire invece su temi delicati che non comprenderebbero direttamente i bambini perché non avrebbero gli strumenti, andando direttamente a enfatizzare quelli che sono i valori che la scuola ci porta e, naturalmente, andando a rafforzare sempre di più quella parte educativa che serve per la crescita della persona, investendo direttamente sul loro futuro. Ecco perché quindi è importante che il Ministero vada ad enfatizzare ancora di più la necessità del coinvolgimento attivo dei genitori all'interno della circolare e ne venga fatta pubblicità tramite i rappresentanti di classe.

recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» (1287). Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*. *(La seduta, sospesa

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'università e della ricerca.

istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato, essa spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Considerato che: le dimissioni sono l'atto con cui un lavoratore dipendente può recedere unilateralmente da un contratto che lo vincola al datore di lavoro; la legge ne subordina l'efficacia al rispetto di una specifica procedura, disciplinata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che consiste nell'impiego di appositi moduli telematici resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a pena di inefficacia, da trasmettere con specifiche modalità al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (cosiddette dimissioni telematiche); considerato inoltre che sono in aumento i casi di lavoratori che si assentano dal lavoro senza alcuna comunicazione per indurre il datore di lavoro ad adottare nei loro confronti un provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata, con il duplice scopo di farsi licenziare ed accedere così alla Naspi; la procedura di licenziamento comporta l'apertura di un procedimento con rilevanti costi, soprattutto per realtà di piccole dimensioni, con ricadute negative di sistema, ammettendo inoltre alla Naspi soggetti che non ne avrebbero diritto; l'articolo 19 del disegno di legge presentato dal Governo, recante «Disposizioni in materia di lavoro» (recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame della 10ª Commissione permanente del Senato) prevede un meccanismo innovativo in materia di risoluzione del rapporto di lavoro; si chiede di sapere quali siano i criteri, la *ratio* e i reali effetti delle disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro contenute nel suddetto disegno di legge governativo. *(Applausi)*. PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, dottoressa Calderone, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti, che mi offrono la possibilità di chiarire la portata applicativa dell'articolo 19 del disegno di legge in materia di lavoro, l'Atto Senato 1264, in tema di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente assegnato all'esame della 10a Commissione del Senato. Come evidenziato dagli interroganti, la Naspi è un'indennità che spetta ai lavoratori a seguito della risoluzione involontaria del rapporto di lavoro. Con l'inserimento del comma 7-*bis* nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, si interviene qualificando correttamente come risoluzione del rapporto di lavoro imputabile a volontà del lavoratore l'assenza ingiustificata, pertanto immotivata, protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni. Il Governo ha inteso colmare una lacuna della normativa in materia di risoluzione involontaria del rapporto di lavoro che, in alcune occasioni, non si è mostrata efficace nel prevenire un utilizzo non corretto della prestazione Naspi, particolarmente nell'ipotesi di mancata giustificazione dell'assenza da parte del lavoratore. Tuttavia, poiché non è interesse del Governo negare le giuste tutele ai lavoratori, la disposizione contempera queste contrapposte esigenze, prevedendo che l'assenza protratta non sia qualificabile come risoluzione volontaria, se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che hanno determinato l'assenza. In un'ottica di semplificazione, vista l'irreperibilità del lavoratore, è prevista inoltre una deroga alla procedura di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che impone la comunicazione in via telematica delle dimissioni. Ancora, in un'ottica di tutela piena ed effettiva, è stabilito l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare l'assenza protratta del lavoratore all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, che potrà verificare la veridicità della comunicazione. Appare evidente, quindi, che la disciplina descritta, pur qualificando come dimissione volontaria l'assenza ingiustificata del lavoratore, presidia però questa fattispecie di una serie di garanzie volte a impedire che tale normativa sia utilizzata in danno del lavoratore. Ritengo dunque sia chiara la *ratio* dell'intervento normativo, che non è assolutamente quella descritta in taluni commenti imprecisi e direi anche frettolosi Non si tratta certamente - lo voglio sottolineare - di dimissioni in bianco. Non è questa la fattispecie e voglio ribadirlo. Con questo intervento abbiamo inteso disciplinare gli effetti dell'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, senza comunque comprimere i diritti e le tutele dei lavoratori.

un ottimo lavoro che sta dando molti frutti, perché si sta intervenendo in maniera efficace su molti aspetti del mondo lavorativo. La domanda era proprio mirata a mettere in risalto la prontezza degli interventi da questo punto di vista. L'immediatezza degli stessi dimostra un'attenzione particolare che viene mostrata da parte del Ministero, nella sua complessità,

*(LSP-PSd'Az)*. Signor Ministro, nei giorni scorsi a Borgo Panigale è avvenuto l'ennesimo incidente. Si è registrato l'ennesimo caso mortale presso lo stabilimento della Toyota, il cui bilancio è di due morti e undici feriti gravi e uno gravissimo. Le autorità hanno disposto il sequestro dell'impianto per agevolare le indagini, portando alla sospensione di tutte le attività produttive e logistiche dello stabilimento. La Toyota ha infatti comunicato la decisione di chiudere lo stabilimento nella zona e fermare tutte le attività lavorative, comprese quelle di *smart working,* e i lavoratori sono stati messi in cassa integrazione dal 23 ottobre. Il 29 ottobre si è svolto un incontro tra la dirigenza e i sindacati per discutere gli ammortizzatori sociali e i sindacati avevano chiesto la cassa integrazione al 100 I rappresentanti dei lavoratori hanno quindi chiesto il completamento della retribuzione e la chiusura a tempo indeterminato agita non poco le 800 persone interessate, ma anche le altre 50 che si trovano nello stabilimento di San Donato Milanese, chiuso anch'esso dopo l'incidente. Le chiedo quindi, signor Ministro, quali ulteriori notizie, fatte salve le indagini della magistratura, può fornire in merito alla causa dell'incidente, affrontando ancora il tema della sicurezza sul lavoro, a fronte anche di quella che abbiamo presentato come la risoluzione che è appena stata votata in quest'Aula. anche quali iniziative intenda prendere di sua competenza per adottare la salvaguardia delle persone coinvolte in questo ennesimo incidente, alla luce anche delle ulteriori informazioni che possono essere emerse nel tavolo tenutosi il 29 ottobre, per assicurare il personale e le famiglie dei due stabilimenti. Soprattutto auspico che questo caso non diventi una scusa e la motivazione per la Toyota per chiudere completamente gli stabilimenti, anche alla luce di quello che sta avvenendo in Germania, che ci preoccupa assolutamente, con la chiusura di tre

sociali*. Presidente, ringrazio la senatrice interrogante e i suoi colleghi per il quesito e l'attenzione dedicata all'incidente che si è verificato qualche giorno fa presso lo stabilimento della Toyota di Borgo Panigale. Voglio prima di ogni cosa esprimere il mio cordoglio e quello del Governo ai familiari delle vittime per questo tragico evento e la vicinanza ai feriti. Quanto accaduto ci impone di mantenere alta l'allerta sui temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per dare un supporto concreto a tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda terribile, lo scorso 29 ottobre ho incontrato, insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, gli esponenti apicali della società Toyota, della Toyota Mondo e della divisione Toyota Italia, i quali mi hanno assicurato che forniranno tutto il supporto necessario ai lavoratori degli stabilimenti coinvolti e alle famiglie delle vittime. L'azienda ha garantito, al fine di non penalizzare il reddito dei lavoratori, che il trattamento di integrazione salariale richiesto per i lavoratori dell'unità interessata dall'incidente, nonché delle unità di Crespellano e di San Donato Milanese, sarà accompagnato da interventi a proprio carico anche mediante anticipazione del trattamento stesso, onde evitare soluzioni di continuità nella percezione della retribuzione durante la temporanea chiusura dello stabilimento, attualmente sottoposto a sequestro penale. Il sequestro in questione interessa anche i *server* aziendali, collocati nella sede di Borgo Panigale, e per questo incide sull'operatività degli ulteriori stabilimenti, per i quali l'azienda ha garantito comunque le massime tutele, che si estendono anche a profili ulteriori quali maturazione delle ferie, dei permessi e della tredicesima mensilità. Sono state fornite dagli stessi vertici della società rassicurazioni circa la prossima trasformazione dei contratti di lavoro dei lavoratori in somministrazione in contratti a tempo indeterminato, nonché l'assunzione a carico dell'azienda di ogni onere e spesa derivanti dall'incidente a favore delle famiglie dei lavoratori coinvolti. Le informazioni fornite trovano ampio riscontro nell'accordo sindacale sottoscritto il 29 ottobre tra le organizzazioni sindacali e i responsabili di Toyota e dello stabilimento interessato dall'incidente. Nel testo dell'accordo sono stati confermati gli impegni assunti con il Ministero ed è stata definita in modo concordato la strategia da adottare per la messa in sicurezza del sito per il riavvio della produzione, anche in riferimento alle prospettive di stabilizzazione dei lavoratori a termine in somministrazione. In ogni caso, i vertici di Toyota hanno chiarito la volontà di mantenere l'operatività dello stabilimento di Bologna e di proseguire l'attività dello stabilimento di Crespellano e di San Donato Milanese.

nei siti produttivi di cui vi ho parlato. Pur non essendo possibile fare anticipazioni, vista l'attività di accertamento in corso da parte dell'autorità giudiziaria, auspico, esprimendo massima fiducia nell'operato delle autorità, che le attività di indagine possano portare presto a esiti che chiariscano la dinamica della vicenda, permettendo la ripresa dei cicli produttivi interrotti a causa dell'incidente che si è verificato nello stabilimento di Borgo Panigale. Sottolineo, per quanto ci riguarda e per quanto ci consta dalle affermazioni e dalle rassicurazioni che abbiamo ottenuto in questo momento, che dobbiamo soltanto accompagnare i lavoratori e l'azienda nella definizione di tutti i percorsi, a tutela ovviamente anche della salute e della sicurezza dei lavoratori. Non c'è però una volontà di disimpegno dell'azienda nei confronti di quelle che invece sono attività produttive assolutamente strategiche, perché lo stabilimento di Borgo Panigale è l'unico, per quanto riguarda la Toyota, che produce i carrelli elevatori che poi vengono utilizzati negli stabilimenti in tutto il mondo. non si può morire di lavoro ancora nel 2024. Questo Governo sta facendo tanto sulla sicurezza sul lavoro, ma purtroppo abbiamo visto che non basta. Anche oggi un operaio nel bergamasco - lo abbiamo ricordato prima

padre. La risoluzione che è stata approvata in Commissione ha proprio il fine non solo di ragionare su prospettive di nuove legislazioni, ma anche di andare direttamente su qualcosa di fatto. Dall'altro punto di vista, le sue parole sono rassicuranti, perché evidenziano quanto impegno vi sia da parte del Governo per assicurare a questi lavoratori, che da un giorno all'altro si sono ritrovati senza lavoro, che si vedranno garantito almeno lo stipendio, coperto al 100 per cento, in vista poi della riapertura dello stabilimento. Sicuramente sono anche rassicurazioni quelle che ci sta dando. dando. Con la crisi dell'*automotive* che si sta verificando a livello europeo, con la decisione di andare verso la transizione ecologica senza una visione, anzi direi senza una transizione industriale e quindi senza una prospettiva, ci poteva supportare la motivazione della chiusura dello stabilimento.

come anche lei ha sottolineato - che è importante lo sportello, perché in questo periodo di transizione è sicuramente rilevante un supporto per la famiglia e per i lavoratori

vorremmo parlare con lei di tante cose, dai dossieraggi di questi giorni a ciò che è accaduto attorno alla piattaforma SDI di pertinenza del Viminale, fino ai misteriosi 65 morti di giugno nel mare di Roccella Ionica, scomparsi dai *radar* e lasciati al dolore silenzioso dei familiari. Potremmo anche parlare dell'aumento dei reati in materia di pubblica sicurezza e dell'annunciato ritiro - punto di domanda da parte del Governo del decreto flussi, da lei enfaticamente - quanto cripticamente, se posso permettermelo - annunciato *urbi et orbi* nel salotto di Vespa, fino allo scontro attualmente in corso nel decreto *cyber*. Tuttavia, il tempo è tiranno e i soldi sono pochi, quindi veniamo all'oggetto della questione, che è relativa alla vicenda che si è realizzata lo scorso 13 ottobre, quando - lei ne è ben cosciente 16 migranti sono stati imbarcati - non si sa da dove - a bordo di una nave della Marina. Quei 16 migranti, di cui due minorenni e altri due che versavano in condizioni di salute precaria - che sono stati prontamente trasferiti in Italia a bordo di navi della Marina militare - hanno fatto parte del famoso pacchetto dei 12 per i quali l'autorità giudiziaria ha disposto il rimpatrio per effetto della mancata convalida dei relativi decreti di trattenimento. Secondo alcune stime indipendenti, il costo del trasferimento in Albania per singolo migrante e per singola tratta è pari a 20.000 euro. Di conseguenza, l'onere sostenuto dall'Italia per i soli trasferimenti di andata e ritorno di quei 16 migranti sarebbe pari a 640.000 euro, senza contare il personale e i mezzi delle Forze dell'ordine impegnati in tali operazioni. Alla luce di ciò, e quindi dovendo valutare l'economicità, l'efficienza e l'impatto economico, siamo a chiederle, anche alla luce del piano strutturale di bilancio e dei tagli che state realizzando sul Dicastero da lei retto, esattamente in quale punto del mare siano stati soccorsi quei 16 migranti, a quale distanza dalla più prossima costa italiana siano stati raccolti e in quali condizioni.

Signor Presidente, premetto che le operazioni di recupero e trasferimento in Albania dei 16 migranti di cui al quesito si sono svolte in acque internazionali, in due distinti eventi avvenuti in zona SAR (search and Tutte le attività sono state condotte nel pieno rispetto di procedure operative standardizzate e definite in precedenza da un tavolo interforze, con il coinvolgimento dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) e dell'agenzia ONU per i rifugiati. Il progetto Albania, sul quale - lo ricordo - abbiamo registrato il forte interesse di 15 Paesi europei e soprattutto della Presidente della Commissione europea, risponde all'obiettivo prioritario del Governo di prevenire e contrastare i flussi migratori irregolari e potrà in futuro svolgere un'importante funzione di deterrenza, con conseguenti benefici che si rifletteranno anche sul lavoro e sui compiti delle Forze di polizia. A mio giudizio, è stata posta una pregiudizievole attenzione rispetto a una singola operazione di recupero e trasferimento di migranti svolta da assetti navali pubblici, se si tiene conto che i numeri delle operazioni di analogo tipo nell'ultimo decennio evidenziano una media di centinaia di interventi all'anno, con punte di arrivi, in determinati periodi, che hanno gravato in maniera eccezionale sugli oneri a carico della finanza pubblica, nonché sul sistema dell'accoglienza. Trattasi di un fardello economico (solo nel 2023 di circa due miliardi di euro), oltre che gestionale, che il Governo in carica ha ereditato da epoche precedenti di rassegnazione e assenza di ogni qualsivoglia reazione agli arrivi massicci e incontrollati. Segnalo inoltre che il costo reale dell'impegno della nave Libra si è rivelato di 8.400 euro complessivi, al netto delle spese di ordinario esercizio quotidiano della nave; un costo giornaliero ampiamente inferiore a quello che veniva sostenuto in epoca di grande celebrazione di operazioni come Mare Nostrum, che richiedevano oneri per 300.000 euro al giorno. In ogni caso, tutte le azioni ad ampio raggio poste in essere da questo Governo contrappongono il forte calo del numero degli arrivi via mare dei migranti: meno 62 per cento rispetto all'anno scorso e meno 30 per cento rispetto al 2022. Con il Governo in carica è finita anche la stagione dei tagli indiscriminati alle politiche di sicurezza e del mancato riconoscimento della specificità e della rilevanza dei compiti svolti dalle Forze di polizia. Rassicuro l'onorevole interrogante sul fatto che il taglio del *turnover*, previsto dal disegno di legge di bilancio per il pubblico impiego in generale, non riguarda le Forze di polizia, proprio in ragione della loro specificità ordinamentale, affermata da altri provvedimenti di questo Governo. Questo Governo, infatti, sin dal suo insediamento ha dedicato importanti risorse a tutto il comparto, a cominciare dal fondo per le assunzioni della legge di bilancio per il 2023, che sta consentendo di ringiovanire e potenziare gli organici. Solo nel 2023 ci sono state 15.000 nuove assunzioni, di cui oltre 3.500 oltre 3.500 in aggiunta al *turnover*. Anche nei recenti provvedimenti finanziari all'esame del Parlamento, a partire dai 100 milioni per lo straordinario delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, sono stati previsti importanti stanziamenti per l'imminente rinnovo contrattuale e investimenti destinati al rafforzamento e all'ammodernamento di mezzi e strutture. Abbiamo sempre avuto e continuiamo ad avere come priorità la sicurezza dei cittadini, dopo anni e Governi precedenti che hanno considerato il sistema sicurezza un fattore di costo e non di investimento; scelta sbagliata e non priva di effetti, che ancora adesso fatichiamo a invertire. Signor Presidente, stupirò il Ministro: mi dichiaro soddisfatto di una parte della sua replica, perché ha detto esattamente quello che noi temevamo, cioè che quei 16 cittadini sono stati raccolti nel mare, in acque internazionali, fra l'Italia e la Tunisia. Ci chiediamo quindi il motivo per il quale, anziché portarli nel primo porto sicuro, Lampedusa, siano stati portati in Albania, aprendo il balletto nel quale siamo e siete ancora tutti immersi. Non voglio neanche inserirmi all'interno di un terreno sdrucciolevole nel quale vedo che si sta

2016. Ad agosto ci sono stati infatti 399 morti e 487 dispersi, con un incremento di persone che non ci sono più nel Mediterraneo del 34 per cento rispetto al 2023. Tutta questa operazione, però, si sta dimostrando totalmente inefficace, perché la legge parla di 670 milioni per l'attuazione del protocollo, a cui vanno aggiunti tanti altri costi nascosti e imprecisati oneri aggiuntivi per il costo del personale, utenze, trasferte, carburante, procedure burocratiche e trasferimenti dei migranti. Solo le 22 aule per le udienze ci sono costate quasi due milioni. Tenete Tenete fermi i poliziotti in questo momento in Albania, con un costo aggiuntivo di 900.000 euro di indennità di trasferta per guardare il nulla; portate i migranti che dovrebbero sbarcare prima in Albania, spendendo di più per farli poi riportare in Italia; nel frattempo, la sicurezza nelle nostre città continua a diminuire, i reati aumentano e la situazione è quella che è dal punto di vista complessivo. Se questo non è un fallimento, signor Ministro, mi dica lei come lo definisce.

*(M5S)*. Signor Ministro, della strage di Roccella Ionica - di cui la storia un giorno le chiederà la verità e sarebbe un bene per tutti, anche per il Governo, se la verità venisse alla luce subito - la trasmissione «Report» nella puntata del 27 ottobre 2024 ha ricostruito le fasi successive al naufragio in cui, nella notte tra il 16 e il 17 giugno 2024, al largo del Mar Ionio, persero la vita 65 persone, tra cui 26 bambini. Dopo l'allarme lanciato da un velista francese, sarebbe seguito l'arrivo di un mercantile inviato dal centro coordinamento soccorso marittimo che ha raccolto i naufraghi, per poi trasportarli sulla motovedetta della Capitaneria di porto partita da Roccella. Ebbene, sembrerebbe che i cadaveri siano arrivati a spezzoni in diverse e distanti zone tra loro al pari dei sopravvissuti, sparpagliati negli ospedali di più Province, e che i Paesi di provenienza delle persone che viaggiavano a bordo di quella maledetta imbarcazione fossero Afghanistan, Iran, Iraq, Siria e Pakistan Paesi devastati da guerre e violazioni dei diritti - e che la rotta fosse la stessa della strage dei migranti allo Steccato di Cutro. È evidente che, anche nel caso in parola, emergono ipotesi di responsabilità per la sottovalutazione da parte delle autorità competenti nell'autorizzazione al soccorso dei naufraghi e per non aver dato corso all'allerta lanciata il 16 giugno 2024 da Alarm Phone al centro coordinamento soccorso marittimo di Roma, della richiesta di aiuto giunta da una barca in difficoltà nello Ionio, dando anche la sua esatta posizione. Risulta altresì da fonti di stampa la fulminea promozione del viceprefetto che si occupava del caso caso ed oggi è assessore regionale e che la comunicazione delle istituzioni sulle operazioni successive al soccorso sia avvenuta per il tramite di brevi comunicati, spesso incompleti e incoerenti. La concatenazione di tutti questi eventi non considerabili più casuali desta gravi preoccupazioni in ordine ad un apparente sistema finalizzato all'occultamento dei fatti e della realtà, ovvero sulla base di una consegna del silenzio. Tutto questo premesso, noi vi chiediamo di sapere se vi sia la volontà politica di non chiarire la dinamica dei fatti occorsi, della loro esatta concatenazione, della disamina degli ordini impartiti, delle responsabilità delle regole d'ingaggio e della catena di comando delle istituzioni coinvolte e se vi sia altresì la volontà politica volontà politica di non chiarire le condotte tenute nei confronti dei giornalisti, nonché dei familiari delle vittime, anche con riguardo agli accordi presi con i familiari stessi e con i loro Paesi di origine per il rientro delle salme.

internazionali, iniziato in un'area SAR non di competenza italiana e rispetto al quale, nonostante tutto, le autorità italiane - lo sottolineo - sono state le prime ad attivarsi e a gestire concretamente le fasi di ricerca e di soccorso. Il Centro di coordinamento delle capitanerie di porto, sin dalla prima segnalazione ricevuta il 16 giugno scorso, si attivava immediatamente per rintracciare l'imbarcazione attraverso una serie di verifiche e controlli tramite le compagnie telefoniche e gli assetti aeronavali di Frontex impegnati nella sorveglianza di quell'area, dirottava una nave mercantile che, giunta in zona, non avvistava alcuna unità in *distress*, trasmetteva a tutte le navi in transito la richiesta di prestare la massima attenzione all'avvistamento di una possibile imbarcazione in difficoltà inviava una motovedetta della Guardia costiera al confine tra la zona SAR italiana e quella greca per il trasbordo delle 12 persone presenti a bordo dell'imbarcazione privata francese che, nel frattempo, era intervenuta nella zona. Dai primi elementi di informazione raccolti in quel frangente è stato ipotizzato che vi fossero circa 70 migranti e quindi si è proceduto senza sosta fino al 25 giugno incluso alla ricerca di eventuali dispersi in mare con l'avvistamento ed il recupero di 35 salme. La prefettura di Reggio Calabria ha sempre dato notizie alla stampa, anche in orario notturno, di tutte le operazioni di recupero e sbarco delle salme sia mediante i comunicati stampa (sono rinvenibili) inviati via *e-mail*, sia mediante una *chat* rivolta a circa 50 giornalisti, realizzando anche un'apposita sezione del proprio sito Internet dedicata al naufragio (basta controllare). Dal 19 giugno è stato inoltre attivato un punto informativo presso il porto di Roccella Ionica, con la presenza di mediatori culturali, per fornire un adeguato supporto psicologico e di assistenza ai parenti delle persone coinvolte nel naufragio. La distribuzione delle salme e il ricovero delle persone sono stati effettuati esclusivamente sulla base delle rispettive disponibilità al momento esistenti. Una considerazione conclusiva a riprova delle imprecisioni contenute nella predetta ricostruzione giornalistica riguarda proprio l'asserita promozione ad assessore regionale di una funzionaria del Ministero dell'interno che in realtà è stata interessata per sua autonoma disponibilità ad una nomina estranea all'amministrazione di appartenenza nella prospettiva di un prossimo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Lei ci ha restituito esattamente le stesse informazioni che noi le abbiamo dato in sede d'interpello, ce le ha ripetute. Noi non le abbiamo chiesto chi è arrivato per primo o tutto quello che risulta dagli atti. Noi le abbiamo chiesto spiegazione del blocco dei giornalisti ai quali non veniva permesso di avvicinarsi ai siti, addirittura nemmeno di entrare negli ospedali per scambiare magari qualche parola con i superstiti. Noi le abbiamo chiesto un chiarimento sulla catena decisionale, le abbiamo chiesto informazioni sulla tutela dei diritti dei familiari, sulla tutela del diritto dell'informazione, sulla tutela del diritto dei giornalisti di venire, osservare, guardare e raccontare. Questa sua risposta, che non fa altro che richiamare dati burocratici ufficiali che sono agli atti - dice bene lei: basta andarli a leggere - non chiarisce nulla, chiarisce solo una cosa: in questo Paese è giusta la preoccupazione per la china illiberale che il Governo ha voluto intraprendere a discapito della democrazia e della libertà.

Signor Presidente, questa interrogazione in pratica è nata a settembre. Era metà settembre quando il ministro Crosetto affermò che in più di un'occasione i Servizi non avevano dato informazioni alla Difesa, cosa che avrebbe potuto creare problemi alla sicurezza del Paese. Un'affermazione enorme, un Ministro della difesa che chiamava in causa i Servizi e quindi il delegato ai Servizi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano.

che ha generato questa interrogazione. È noto quello che è successo: il sistema di indagine dello stesso Ministero da lei guidato è stato violato. Sono stati interrogati 800.000 dati SDI e il regista sarebbe stata la società Equalize di Milano, di proprietà di Enrico Pazzali, Presidente della Fondazione della Fiera di Milano. Le dimensioni del sistema violato sono impressionanti. Il pubblico ministero Francesco De Tommasi della Direzione distrettuale antimafia ha parlato di creazione di vere e proprie banche dati dati parallele vietate, di indagati pericolosissimi e di appoggi ad alto livello e a vari ambienti, anche quello della criminalità mafiosa e dei servizi segreti, pure stranieri. Abbiamo letto di contatti con qualche agente del Mossad, per dire. Ci sono state informazioni sensibili anche dirottate verso l'estero. Per questo noi siamo allarmati, Ministro, e chiediamo al Governo di capire cosa è successo perché quest'attività di spionaggio, che ha violato le banche dati del nostro Paese che contengono dati molto sensibili, ha riguardato la finanza, l'impresa, la politica, la seconda carica dello Stato e perfino un indirizzo di posta elettronica del Presidente della Repubblica. Quindi, chiediamo di sapere quanto è a rischio la sicurezza del Paese e cosa state facendo per tutelare la cybersicurezza da ingerenze della criminalità e di potenziali servizi stranieri. Perché avete rinviato il Consiglio dei Ministri? Quali contrasti ci sono? Fateli sapere al Paese e al Parlamento.

accertare il quadro delle responsabilità e il reale perimetro di attività e di interesse degli indagati. Il quadro degli illeciti che emerge al momento è preoccupante e impone a tutti gli attori del sistema di sicurezza di effettuare ogni accertamento e ogni approfondimento pertanto immediatamente incaricato il Capo della Polizia di avviare le conseguenti verifiche interne sulla sussistenza di ipotizzati accessi abusivi alle banche dati del Viminale e in particolare del CED Interforze, o sull'utilizzo illecito delle stesse. All'esito dei primi controlli, l'ipotesi di compromissione delle infrastrutture del CED del Ministero dell'interno da remoto non è risultata allo stato riscontrata, ferme restando le attività investigative in corso. Su questi comportamenti, ove accertati, il Governo e il Ministero dell'interno saranno estremamente severi. La stessa severità sarà riservata anche a coloro i quali dovessero risultare responsabili di comportamenti omissivi rispetto ai compiti di controllo e vigilanza già previsti dalle attuali regole di sicurezza. Ricordo che lo scorso dicembre avevo già dato mandato al Capo della polizia di procedere all'aggiornamento della commissione tecnica, non operativa da decenni, incaricata per legge di analisi costanti per garantire *standard* sempre più elevati nella gestione delle informazioni sensibili. Abbiamo dunque già avviato i lavori per l'implementazione e il potenziamento del livello di sicurezza del sistema attraverso la definizione di criteri e misure tecniche più stringenti per l'accesso al CED Interforze. Il costante impegno sul versante della sicurezza informatica trova ulteriore conferma nell'aver dato concretezza, dallo scorso febbraio, al servizio per la sicurezza cibernetica nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, presso cui operano specialisti che curano le attività inerenti alla sicurezza delle reti dei sistemi informativi e delle infrastrutture informatiche in uso al Ministero dell'interno, in linea con i più aggiornati *standard* previsti a livello internazionale. Le indagini condotte dalla procura di Milano, dalle quali emerge che i reati di cui trattasi sono stati commessi anche nel 2021 e 2022, richiamano il complesso e delicato tema della tutela *cyber* delle istituzioni e il Governo, fin dal suo insediamento, ha evidenziato una forte sensibilità al tema, come dimostra la prima legge organica in materia di prevenzione e contrasto al crimine informatico e di rafforzamento complessivo della cybersicurezza nazionale approvato con la legge 28 giugno 2024, Nel contesto di un mirato inasprimento del quadro sanzionatorio penale per i reati informatici più gravi, è stato anche rimodulato il reato di estorsione, adattandolo alle dinamiche dei programmi informatici dannosi che compromettono i dispositivi digitali a fini di riscatto, il cosiddetto *ransomware*. Segnalo, infine, che per il potenziamento delle reti dei servizi e dei sistemi *cyber* della pubblica amministrazione, abbiamo finanziato con oltre 715 milioni di euro specifiche progettualità che saranno sottoposte ad azione di monitoraggio. Signor Ministro, non siamo soddisfatti della risposta. Io non nego che lei, nel suo ambito, nel suo Ministero, faccia quello che deve fare; qualcosa ha ereditato, ma noi siamo preoccupati in generale, per questo abbiamo chiamato in causa la Presidente del Consiglio, sia per quelle frasi del suo Ministro della difesa che interloquiva, lo dico tra parentesi, con il Sottosegretario delegato ai servizi, sia perché - lei richiamava il 2021 - l'allora ministro dell'innovazione Colao parlò ufficialmente dicendo che le banche dati pubbliche per il 90 per cento non avevano gli *standard* minimi di sicurezza. Siamo in tempi di guerra, siamo in tempi di aggressione economica e finanziaria. Il nostro è un Paese vulnerabile da molti punti di vista, compreso quello della cybersicurezza. Ci aspettiamo, Ministro, che se ne faccia interprete e lo dica alla sua Presidente del Consiglio che su temi come questi (la sicurezza nazionale) si venga con trasparenza in Parlamento e si dica quanto ha rischiato e quanto rischia il Paese e che cosa si può fare. Si coinvolgano le opposizioni su temi come questi. Non si può uscire dal *bunker* di Colle Oppio per andare al *bunker* di Palazzo Chigi con l'elmetto. La si smetta con le teorie del complotto. Tra l'altro a Milano, se proprio si vuole dire questo, sembra proprio esserci un complotto interno alla destra. Noi non abbiamo chiamato in antimafia la destra milanese per capire cosa c'è stato dietro, quali complotti, quali guerre, non è questo il punto. A noi interessa la sicurezza del Paese che è a rischio e chiediamo che il Governo, con trasparenza, davanti al Parlamento, dica cosa si può davvero fare, perché in un momento come questo l'Italia dev'essere protetta. La vulnerabilità del Paese è un interesse nazionale e noi siamo disposti - ma se farete sul serio - a collaborare. Mi pare però che sul serio non stiate facendo.

dell'interno* - Premesso che: la recente indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano avrebbe rilevato l'esistenza di un sodalizio criminale che, attraverso una serie di accessi illeciti ai sistemi d'indagine delle forze dell'ordine e a banche dati pubbliche, avrebbe posto in essere un'ampia attività di dossieraggio di cittadini, esponenti delle istituzioni, imprenditori e professionisti; al centro dell'indagine vi è la società Equalize S.r.l., attualmente sotto sequestro, che avrebbe creato un sistema per accedere illegalmente a dati sensibili per poi vendere le informazioni acquisite illecitamente; tra gli indagati vi sono il presidente di fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali e l'ex poliziotto Carmine Gallo, entrambi soci della società; le notizie riportate dalla stampa restituiscono un quadro allarmante che sollecita interventi a tutela delle banche dati pubbliche e dei dati personali e sensibili dei cittadini; la recente legge 28 giugno 2024, n. 90, ha disposto un inasprimento del quadro delle sanzioni previste per i reati informatici e l'aumento degli standard di sicurezza informatica degli enti pubblici e privati, prevedendo, a tal fine, il potenziamento delle misure di protezione e prevenzione per contrastare le minacce del cyber crimine sempre più sofisticate, si chiede di sapere quali quali ulteriori iniziative intenda adottare il Governo per rafforzare la sicurezza delle banche dati pubbliche e, in particolare di quella del Ministero dell'interno, al fine di prevenire il ripetersi di simili, gravi episodi, e per assicurare elevati livelli di protezione delle infrastrutture critiche del nostro Paese.

Il Ministero dell'interno ha intrapreso da tempo un percorso di valutazione e di miglioramento per garantire *standard* elevati nella gestione delle informazioni sensibili, fermo restando che le banche dati del Viminale presentano, dal punto di vista tecnologico, adeguati livelli di sicurezza. Aggiungo che, in relazione allo stato attuale delle indagini, la prefettura di Milano, lo scorso 28 ottobre, ha provveduto a sospendere le licenze concesse in favore di due indagati per l'esercizio di attività investigativa privata e di raccolta di informazioni commerciali. Le indagini di Milano, ma anche quelle che nel recente passato hanno evidenziato attività illecite finalizzate al dossieraggio, pongono il tema della gravità dei comportamenti di chi potrebbe utilizzare dati illecitamente acquisiti, non solo per scopo di lucro, ma anche per attaccare gli avversari politici, alterando le regole della democrazia. È indubitabile che il Governo, sin dal suo insediamento e quindi ben prima delle indagini a cui ho fatto cenno, abbia riservato una specifica attenzione al potenziamento della sicurezza cibernetica. Ne costituiscono prova prova evidente il lavoro sul piano organizzativo delle strutture dedicate, a partire dall'Agenzia per la sicurezza cibernetica, e sul piano normativo l'approvazione della recente legge n. 90 del 2024. Con tale legge è stata prevista un'articolata serie di interventi che vanno proprio nella direzione di implementare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei crimini informatici e di rafforzamento complessivo della cybersicurezza nazionale. Nel contesto di un mirato inasprimento del quadro sanzionatorio penale per i reati informatici più gravi, è stato anche rimodulato il reato di estorsione adattandolo alle dinamiche dei programmi informatici dannosi che compromettono i dispositivi digitali a fini di riscatto (il cosiddetto *ransomware*). Un particolare approfondimento è stato svolto in relazione ai legami tra la sicurezza informatica e quella economico-finanziaria, prevedendo una configurazione del Nucleo per la cybersicurezza, a cui partecipano il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e il governatore della Banca d'Italia, che appena due giorni fa si è riunito per approfondire ed affrontare in chiave sistemica i più attuali attuali aspetti legati alla sicurezza informatica del Paese. Le capacità di prevenzione e risposta della minaccia cibernetica attribuite alla Polizia postale sono state ulteriormente implementate mediante la creazione di appositi nuclei operativi coordinati dal Centro nazionale anticrimine informatico e per la protezione delle infrastrutture critiche, in grado di gestire tra il 2022 e il 2023 oltre 25.000 attacchi informatici classificati come rilevanti e più di 8.000 nei primi otto mesi del 2024, nonché attraverso la costituzione di un'apposita sezione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo dedicata proprio alla minaccia *cyber.* Ministro, lei ci ha ricordato quanto, da un anno a questa parte, è stato fatto per difendere le nostre infrastrutture telematiche e i nostri servizi di sicurezza. D'altra parte, in quest'Aula il 19 giugno abbiamo approvato il disegno di legge sulla cybersicurezza e il Parlamento, nei termini che ci erano stati dettati dall'Unione europea, ha adottato la direttiva NIS2, che cerca di mettere in sicurezza le banche dati pubbliche e anche quelle private, creando un sistema resiliente per aiutare imprese e pubblica amministrazione a difendersi da questi attacchi. Siamo certi che si stia andando nella giusta direzione. Lei ci ha detto che il Governo non è fermo da questo punto di vista, ma è impegnato ad adottare ulteriori sistemi di difesa cibernetica. Pertanto le dico, a nome del sottoscritto e del Gruppo che in questo momento mi onoro di rappresentare, ci dichiariamo soddisfatti della sua risposta.

magistrale in medicina e chirurgia in odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Il provvedimento delega il Governo ad attuare una riforma di sistema volta a garantire un'offerta universitaria di eccellenza e conseguentemente a potenziare il nostro sistema sanitario nazionale in termini di fabbisogno di professionisti. La nuova disciplina sostituirà l'attuale modalità di accesso basata sul *test* unico nazionale, introducendo un modello originale fondato su un percorso di studi comune che consentirà allo studente meritevole di essere indirizzato verso il percorso formativo a lui più consono. le chiediamo di sapere quali ulteriori obiettivi strategici, oltre a quelli già indicati, si intenda conseguire con tale riforma e in che modo si intenda incentivare le studentesse e gli studenti ad optare per i percorsi meritocratici istituiti nell'ambito delle università italiane.

proprio qui in Senato, come ricordava il senatore Occhiuto, è partito l'*iter* del disegno di legge che delega il Governo, e quindi il Ministero che mi onoro di servire, a rivedere i criteri di accesso ai corsi di laurea in discipline mediche. È un percorso che abbiamo iniziato due anni fa e che ora raggiunge una tappa fondamentale. Voglio ancora una volta ringraziare il presidente Marti e il presidente Zaffini, che seguirà il provvedimento anche nel suo passaggio in Aula come relatore, tutti i senatori della 7a Commissione istruzione per il prezioso lavoro di questi mesi; una collaborazione fatta di ascolto, valutazioni, ma soprattutto di scelte condivise, che si è poi concretizzata nel testo unificato, frutto della mediazione di tutte le forze politiche. I senatori hanno lavorato con grande competenza e con impegno, anche per sottrarre un argomento così importante per le nostre studentesse, per i nostri studenti e ancor più in generale per il Paese ancor più in generale per il Paese a un arido scontro tra opposte tifoserie, tra difensori dell'accesso a numero chiuso con *test* d'ingresso e sostenitori dell'accesso liberissimo. La modalità d'ingresso prevista dal testo della riforma propone un percorso aperto, sostenibile e progressivo. Come lei ha correttamente sottolineato, senatore Occhiuto, si tratta di un modello italiano, che non è mutuatario, soprattutto in termini di tempo, di alcunché dal modello francese, dove la selezione verrà effettuata solo a seguito di un'adeguata preparazione svolta dalle università. Gli aspiranti medici si prepareranno non più per fare *test*, ma studiando materie caratterizzanti. Stiamo lavorando su un tempo congruo per valutare le competenze acquisite; vogliamo verificare non solo il merito, ma anche la reale attitudine dei futuri medici a proseguire lungo un percorso di formazione che è anche una missione di vita. Con questa riforma - lei lo ha ricordato - eliminiamo quello sbarramento troppo casuale fatto di *test* a crocette, che ha costretto troppi studenti a recarsi in altri Paesi della Comunità europea, con conseguente sacrificio economico e con un livello qualitativo molto spesso nettamente inferiore dell'offerta formativa. Vogliamo dire basta - questo è il nostro obiettivo strategico - a medici con cittadinanza italiana che si sono laureati all'estero in un Paese UE, come vengono comunemente definiti i nostri studenti che acquisiscono il titolo all'estero. Vogliamo medici cittadini italiani laureati in Italia. Dirò di più. Dobbiamo creare le condizioni - questo è un altro obiettivo strategico perché i ragazzi che sono stati costretti ad andare a studiare all'estero possano rientrare nel nostro Paese. Ci tengo però a ricordare che nulla andrà perso. Chi non avrà un bilancio finale sufficiente a consentire da subito l'immatricolazione al corso prescelto potrà comunque reinvestire le conoscenze e le competenze acquisite in un altro percorso formativo contiguo, senza sprecare tempo e risorse. Per evitare i danni del domani occorre lavorare sull'oggi e per questo dobbiamo rendere le nostre università più attrattive rispetto a quelle estere e ancora di più all'altezza di soddisfare le richieste del nostro sistema sanitario, formando medici competenti, motivati, appassionati e in numero sufficiente. nuova finestra") *(FI-BP-PPE)*. Signor Ministro, la ringrazio per la risposta puntuale, che mi soddisfa e che soddisfa l'obiettivo della riorganizzazione del sistema delle professioni medico-sanitarie; un obiettivo che va portato avanti in un'ottica di programmazione e, allo stesso tempo, di sostenibilità, sia per gli atenei che per il Servizio sanitario nazionale, puntando a garantire il fabbisogno di medici negli anni a venire. L'intento è quello di garantire una selezione più equa, che sia basata però sulle competenze acquisite dagli studenti. A regolare l'accesso saranno infatti i crediti formativi e la posizione raggiunta in una graduatoria nazionale. Si aggiunga a questo che la sua riforma prevede anche iniziative di orientamento per i ragazzi della scuola secondaria ci saranno anche percorsi specifici per favorire l'ingresso nei corsi di laurea, garantendo a tutti i ragazzi che lo meritino la possibilità di diventare professionisti in ambito medico. Quindi la ringraziamo, Ministro, soprattutto per il coraggio con cui ha scritto questa importante riforma degli accessi alla facoltà di medicina, che è attesa da molti ragazzi e da molte famiglie, da tanti anni.

ed altri Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (1287) previ Grazie